"Il link apre una nuova finestra"). Comunico che, in data 17 marzo 2023, è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione

e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech»

20 dicembre 1993, n. 533, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Lazio a seguito del decesso del senatore Bruno Astorre (ricordo che nel pomeriggio lo ricorderemo in quest'Aula), ha riscontrato, nella seduta odierna, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista è Filippo Sensi. Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatore Filippo Sensi. Benvenuto. Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali ricorsi.

Signor Presidente, onorevoli senatori, il prossimo Consiglio europeo, che è il terzo dal giuramento del Governo, ha nella sua agenda sfide prioritarie per l'Unione europea, sfide che sono state anche al centro del dibattito dell'ultimo Consiglio europeo straordinario lo scorso 9-10 febbraio: l'Ucraina, la competitività, il mercato unico, l'economia, l'energia, l'emigrazione. In questa fase complessa per il sistema internazionale, l'Unione europea è probabilmente chiamata al compito più arduo degli ultimi decenni: garantire la sicurezza del nostro Continente di fronte alla minaccia rappresentata dalla guerra di aggressione russa verso l'Ucraina; proteggere e sostenere il nostro tessuto socio-economico rispetto all'impatto che da quella aggressione deriva; predisporsi ai cambiamenti radicali che potrebbero profilarsi negli equilibri globali. Tutto questo ovviamente nel rispetto e nel sostegno dei valori di democrazia e libertà che ispirano il nostro percorso, ma che questo tempo necessariamente ci ha insegnato, una volta di più, a non dare necessariamente per scontati. L'Europa e l'intero Occidente sono chiamati a rispondere a questa grande sfida con visione, strategia, efficacia e tempestività. l'Italia, che ho l'onore di rappresentare nel Consiglio europeo, ha oggi tutte le carte in regola per recitare in Europa un ruolo da protagonista e non da comprimaria. È esattamente quello che intendiamo fare, forti della nostra storia, della nostra collocazione geostrategica, della stabilità delle nostre istituzioni e del nostro Governo e della forza delle nostre idee. Un primo banco di prova è certamente rappresentato dal tema dell'immigrazione, a cui il nostro Governo ha ottenuto che venisse dedicata gran parte della riunione del Consiglio straordinario di febbraio. Noi siamo di fronte a un'emergenza che potrebbe diventare - e sta diventando - strutturale. Questa definizione, che potrebbe sembrare un ossimoro, è invece la più realistica fotografia del contesto che attualmente ci circonda. Alla frontiera meridionale marittima dell'Europa stiamo assistendo a una pressione migratoria senza precedenti e anche la rotta marittima orientale, sebbene con numeri che sono oggi più contenuti, non è meno complicata da gestire, come ben dimostra Come voi sapete, all'indomani di questa disgrazia, ho scritto al Presidente della Commissione europea, al Presidente del Consiglio europeo, al Presidente di turno dell'Unione europea e agli altri *leader* europei per ribadire che noi non possiamo attendere oltre. Non possiamo aspettare inermi il prossimo naufragio, che è inevitabilmente un pericolo insito nei viaggi organizzati da criminali e scafisti senza scrupoli. Le frontiere marittime dell'Italia sono frontiere dell'Europa l'Europa è chiamata a difendere quelle frontiere, perché la posta in gioco sono la vita e la dignità di tantissimi esseri umani, vittime di una tratta ignobile, e allo stesso tempo la sicurezza dell'intero continente. Noi siamo di fronte ad organizzazioni criminali che lucrano sugli esseri umani e vogliamo contrastare con forza questo traffico, come dimostrano i provvedimenti che abbiamo preso proprio in un Consiglio dei ministri che si è svolto a Cutro negli scorsi giorni. Fermare le partenze, collaborare con i principali Paesi di origine e transito dei migranti, aumentare i rimpatri, rendere efficienti i percorsi per la migrazione legale e la protezione umanitaria, dedicare risorse finanziarie che siano adeguate a questi obiettivi; sono queste le priorità che ci siamo dati e sono anche le priorità che abbiamo portato al tavolo dei *leader* europei. Un ruolo chiave dovrà quindi averlo il rafforzamento della collaborazione con i principali Paesi di origine e di transito dei migranti, con risorse finanziarie adeguate agli obiettivi da raggiungere. in quest'Aula abbiamo richiamato la risposta europea alla crisi migratoria del 2015 e l'onerosissimo accordo che ne derivò con la Turchia perché collaborasse a frenare i flussi lungo la rotta balcanica. Ecco io ritengo che pari attenzione e adeguati stanziamenti debbano oggi essere dedicati a contrastare i flussi irregolari lungo le rotte del Mediterraneo centrale e a creare nei Paesi di partenza alternative concrete alle migrazioni in termini di formazione, lavoro e sviluppo economico. Voglio infatti ribadire ancora una volta che prima di ogni ipotetico diritto a migrare, ogni essere umano ha il diritto di non essere costretto a migrare in cerca di una vita migliore. Questo è esattamente l'aspetto che Europa e Occidente hanno, a nostro avviso, in questi anni colpevolmente trascurato. Non solo; per lungo tempo - spesso è accaduto anche a Governi precedenti - l'Italia è stata rimproverata di non fare abbastanza per contrastare i cosiddetti movimenti secondari, cioè gli spostamenti di immigrati irregolari da uno Stato all'altro dell'Unione europea. Al Consiglio europeo di febbraio noi abbiamo lavorato per ribaltare questa prospettiva secondo un ragionamento semplice e logico e, cioè, che c'è un modo solo per fermare i movimenti secondari ed è fermare, a monte, i movimenti primari *(Applausi)* e, quindi, le partenze irregolari. Questo ragionamento comincia finalmente a fare breccia tra i nostri *partner* ed è per questo che io credo sia il momento di spingere con forza su un nuovo modello di gestione delle frontiere esterne, in particolar modo di quelle marittime, la cui specificità è stata finalmente riconosciuta grazie al lavoro e all'insistenza del Governo italiano. È frutto di questa stessa azione politica e diplomatica, recepita nelle conclusioni dell'ultimo Consiglio, la presentazione da parte della Commissione europea di un nuovo piano pluriennale di gestione delle frontiere esterne, con particolare attenzione proprio al Mediterraneo centrale. Il piano contiene affermazioni importanti, probabilmente impensabili fino a qualche mese fa, che sono state tradotte in una comunicazione e in una raccomandazione. La comunicazione ha l'obiettivo di assicurare un quadro rafforzato di sorveglianza e controllo delle frontiere esterne dell'Unione attraverso un pieno ed efficace dispiegamento delle risorse operative di Frontex. È una scelta che io considero condivisibile, che fa finalmente giustizia dei tentativi di alcune famiglie politiche europee di indebolire e snaturare il mandato di Frontex. Il piano pone anche, per la prima volta in maniera compiuta, il principio del coinvolgimento degli Stati di bandiera delle navi ONG nelle operazioni SAR, che non possono e non devono più gravare esclusivamente sugli Stati di approdo. Gli Stati di bandiera, che finanziano le organizzazioni non governative, devono assumersi le responsabilità *(Applausi)* che il diritto del mare attribuisce loro. La raccomandazione invece ha l'obiettivo di portare in tempi rapidi al mutuo riconoscimento, tra i 27 Stati membri, dei provvedimenti di espulsione degli immigrati irregolari, in modo che un ordine di allontanamento emesso dalle autorità italiane sia riconosciuto valido anche negli altri Stati e viceversa. Questa impostazione, unita - come dicevo - al rafforzamento del ruolo di Frontex nel supportare gli Stati membri, vorrebbe portare a rendere finalmente effettive le procedure di rimpatrio degli irregolari: un tema che noi abbiamo posto con forza e che sta molto a cuore al Governo italiano. Sono certamente tutti passi che vanno nella giusta direzione e che segnano un cambio di paradigma rispetto alla narrazione che abbiamo conosciuto finora, ma voglio dire che non possiamo ancora dirci soddisfatti. Nel prossimo Consiglio europeo, la Presidenza svedese e la Commissione europea presenteranno lo stato di attuazione delle misure decise cinque settimane fa, tra cui alcune di quelle che ho citato, l'Italia in quella sede intende ribadire che non c'è più un solo minuto da perdere. *(Applausi)*. Questo è il momento di agire: è ora di tradurre in fatti concreti quelle soluzioni, sulle quali il Consiglio europeo ha lavorato e ha trovato un accordo. Intendiamo vigilare affinché questo processo sia effettivo, rapido e incisivo, perché non vogliamo più piangere vittime innocenti nel Mediterraneo, perché non vogliamo più accettare che la selezione all'ingresso dell'Italia e dell'Europa la facciano gli scafisti e le mafie che li gestiscono perché vogliamo un'immigrazione legale, regolamentata e compatibile e perché l'immigrazione illegale di massa penalizza soprattutto chi, scappando davvero dalla guerra e dalla violenza, avrebbe diritto alla protezione internazionale e spesso non trova aiuto, perché le quote di immigrazione possibile sono coperte da chi arriva illegalmente. Di fronte a questa urgenza sono certa di avere con me la maggioranza degli italiani e mi auguro di avere con me anche la più ampia rappresentanza possibile delle forze parlamentari, anche di opposizione la battaglia politica, per chi ha idee credibili, si può efficacemente condurre senza dover dipingere il proprio avversario come un mostro. Anche nella più feroce polemica politica c'è, a mio avviso, un limite che non dovrebbe mai essere oltrepassato, il limite oltre il quale, per colpire un avversario, si mette in cattiva luce la Nazione intera

perché da sola l'Italia si sta caricando un peso e una responsabilità, che dovrebbero essere condivisi anche da altri *(Applausi)*. Alla fine addirittura si finisce con il danneggiare danneggiare la posizione negoziale dell'Italia sui tavoli internazionali. *(Applausi)*. Lo dico da persona che non ha mai fatto mancare le proprie parole forti e la propria opposizione serrata ai Governi che mi hanno preceduto. criticate ferocemente il Governo, criticate ferocemente me, le scelte che facciamo, i provvedimenti che prendiamo, le nostre eventuali mancanze, ma vi prego: fermatevi un secondo prima di danneggiare l'Italia perché questo fa la differenza.

fronti, compresi alcuni richiami che sono stati fatti e alcune attenzioni che sono state raccontate, sul ruolo che il conflitto in Ucraina può assumere nella destabilizzazione anche del Continente africano. Credo invece che queste siano valutazioni sulle quali bisogna avere concentrazione e attenzione, perché abbiamo già visto come, a volte, i flussi migratori siano stati utilizzati come uno strumento di ricatto geopolitico: penso a quello che accadeva ai confini tra Polonia e Bielorussia, soltanto poche settimane prima dell'aggressione quindi che la particolare situazione geopolitica nella quale ci troviamo richieda un approccio molto approfondito alle materie che stiamo seguendo,

la propria terra; esso sta difendendo anche i valori di libertà e di democrazia sui quali si fonda la nostra civiltà, sui quali si fonda lo stesso progetto europeo. Sta difendendo le fondamenta stesse del diritto internazionale, senza il quale sostituiremmo la forza del diritto il diritto del più forte: non esattamente una buona notizia, neanche per noi. Pochi giorni dopo l'ultimo Consiglio europeo, come sapete, ho testimoniato personalmente, con la mia presenza a Kiev, il pieno sostegno italiano all'Ucraina e alla sua popolazione, in coerenza con l'impegno dell'Unione europea, della NATO e delle altre Nazioni vicine e affini. Un sostegno che sarà assicurato in ogni ambito: politico, umanitario, civile, militare e finché sarà necessario, in coordinamento con i nostri *partner* e con i nostri alleati. Continueremo a farlo senza badare all'impatto che queste scelte possono avere nel breve periodo sul gradimento, sul consenso della sottoscritta, del Governo, delle forze politiche di maggioranza. Continueremo a farlo semplicemente perché è giusto farlo sul piano dei valori e su quello della difesa dell'interesse nazionale. L'aiuto militare all'Ucraina è necessario per garantire la legittima difesa di una Nazione aggredita, in linea con la Carta delle Nazioni Unite. Abbiamo formalizzato un sesto pacchetto di aiuti con misure che rafforzano soprattutto le difese aeree. Che significa, signori? Proteggere la vita dei civili. Significa fornire uno scudo di fronte ai bombardamenti indiscriminati che attaccano infrastrutture vitali per la popolazione, sperando che il popolo ucraino si pieghi dopo essere stato privato di acqua, di luce o di riscaldamento. In questo quadro voglio dire con franchezza che considero puerile la propaganda di chi racconta che l'Italia starebbe spendendo soldi per mandare armamenti in Ucraina sottraendoli di fatto alle tante necessità dei nostri concittadini. Questo è falso, e in quest'Aula lo sappiamo tutti. *(Applausi)*. L'Italia sta inviando all'Ucraina materiali e componenti già in suo possesso, che, per fortuna, noi non abbiamo necessità di utilizzare e che inviamo agli ucraini anche per prevenire la possibilità di doverli un giorno utilizzare noi. Infatti noi inviamo armi all'Ucraina anche per poter tenere la guerra lontana dal resto d'Europa e da casa nostra. Dunque, raccontare agli italiani che se non fornissimo le armi all'Ucraina si potrebbero aumentare le pensioni o si potrebbero tagliare le tasse

Dico di più. Questo Governo, che, come sapete, è abituato a fare tutto ciò che considera giusto per difendere l'interesse nazionale dell'Italia,

come del resto hanno fatto i Governi precedenti un po' di soppiatto, senza, cioè, avere il coraggio di metterci la faccia. Noi crediamo, invece, che su queste cose si debba mettere la faccia non abbiamo paura di dire che rispettare gli impegni assunti è vitale per la nostra credibilità internazionale e per la nostra stessa sovranità nazionale, perché banalmente la libertà ha un prezzo e, se non sei in grado di difenderti, qualcun altro lo farà per te, ma non lo farà gratuitamente. Imporrà i suoi interessi anche a discapito dei tuoi, e non mi pare sia mai stato un grande affare per nessuno. Sul piano geopolitico e diplomatico, le pressioni esercitate su Mosca dal nostro punto di vista sono fondamentali per assicurare il rispetto del diritto internazionale, ma lo sono ancora di più per creare le condizioni migliori per l'avvio di un percorso negoziale per il raggiungimento di una pace giusta; condizioni che finora non sono maturate, ma che dobbiamo ancora perseguire con tenacia, come stiamo facendo ogni giorno. L'aggressione russa ha avuto anche ripercussioni sulla sicurezza alimentare globale, contribuendo alla fragilità dello scacchiere africano e mediterraneo, quindi anche ai flussi migratori illegali. Ribadisco pertanto che sosteniamo l'accordo sull'*export* di grano nel mar Nero che è appena stato rinnovato e crediamo sia centrale anche il tema della futura ricostruzione dell'Ucraina, sulla quale credo che il sistema Italia sia pronto a dare il suo contributo. A questo obiettivo lavoriamo anche con la conferenza sulla ricostruzione che ospiteremo proprio a Roma il prossimo 26 aprile. Naturalmente la situazione che stiamo vivendo ha un impatto molto forte anche sui temi economici che verranno affrontati nel Consiglio europeo di giovedì e venerdì prossimi. Rimane fondamentale l'obiettivo del rafforzamento della competitività e della produttività dell'economia europea, in stretta relazione con la doppia transizione digitale ed ecologica. Su quest'ultima vorrei fare un passaggio e provare a essere ancora una volta chiara. In questa fase geopolitica internazionale non ci sono soluzioni semplici.

ci opponiamo a proposte come il regolamento sulle emissioni di anidride carbonica delle auto o la revisione della direttiva per l'efficientamento energetico degli edifici, perché, così come concepite, si traducono in una penalizzazione dei nostri cittadini e delle nostre imprese e rischiano di esporci a nuove dipendenze strategiche, proprio quando stanno andando in porto gli sforzi per liberarci dalla dipendenza dal gas russo. Sul tema delle dipendenze la Commissione ha presentato proprio in questi giorni un piano articolato e ambizioso sulle materie prime critiche, che si pone l'obiettivo di ridurre la dipendenza europea, particolarmente dalla Cina, diversificando i fornitori e rilanciando le capacità estrattive proprie. Il commissario Breton, nel presentare il piano, ha dichiarato che in Europa abbiamo il 30-40 per cento di quasi la totalità dei minerali necessari al nostro fabbisogno interno ed evidentemente è arrivato il momento di dare i mezzi per estrarli e non accettare più che in Europa si consumi e basta, lasciando la produzione agli altri. Sono parole che sottoscrivo dalla prima all'ultima. Non intendo soffermarmi e non mi soffermerò sul ritardo con cui l'Unione europea approccia questo tema dopo decenni in cui ha rinunciato a questa visione, finendo per consegnarsi a nuove dipendenze, il cui prezzo rischiamo di pagare in questi e nei prossimi mesi; né mi soffermo sul fatto che finalmente si arrivi a queste soluzioni dopo anni nei quali chi sottolineava che ci fosse questa necessità veniva, nella migliore delle ipotesi, definito come autarchico. Vorrei invece dire che il Governo italiano è pronto a fare la sua parte; è assolutamente convinto di dover fare la sua parte e che anche in questo caso un piano di tale ambizione necessita di un quadro finanziario e politico che sia chiaro e coerente. Sul piano finanziario è anche in questo caso necessario comprendere come finanziare queste misure con strumenti che ancora una volta non dovranno limitarsi solo a una maggiore flessibilità sugli aiuti di Stato, mentre sul piano politico questa ambizione chiama in causa gli stessi tempi e i modi della nostra duplice transizione: quanto più questa si accelera con *target* spesso di difficile raggiungimento, in assenza della necessaria diversificazione delle forniture, tanto più si aumenta la nostra dipendenza verso fornitori che oggi detengono quasi un monopolio sulle risorse necessarie ad alimentare la nostra transizione. Porre questi problemi, come stiamo cercando di fare in queste settimane su alcuni importanti *dossier* del *green deal*, non vuol dire certo rinunciare agli obiettivi della sostenibilità ambientale; vuol dire invece rendere quegli obiettivi compatibili con la sostenibilità economica e sociale, da un lato, e con la piena sovranità politica ed economica, dall'altro lato. In questo contesto, la strategia commerciale dell'Unione europea deve tenere in debita considerazione anche concetti come *nearshoring* e *friendshoring*, vale a dire la rilocalizzazione di produzioni nei Paesi vicini o nei Paesi amici. È essenziale mantenere un approccio di ampio respiro e un pieno sostegno europeo che garantiscano parità di condizioni e pieno funzionamento del mercato unico. Questa priorità è ancor più valida anche alla luce del nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, che non deve creare disparità e deve prevedere aiuti circoscritti e temporanei. Anche il completamento dell'Unione del mercato dei capitali costituisce parte integrante della nostra risposta comune. Un mercato dei capitali europei integrato è fondamentale per facilitare gli investimenti privati e colmare le lacune di finanziamento della transizione verde e della transizione digitale. Le conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo riconoscono, grazie anche all'impulso italiano, l'importanza della flessibilità sui fondi europei esistenti. È essenziale anche qui mantenere l'attenzione politica sull'attuazione concreta di queste priorità, a maggior ragione perché non c'è ancora consenso tra i ventisette Stati membri su una strategia a lungo termine di sostegno finanziario europeo alla competitività nella forma di un fondo per la sovranità europea volto a sostenere gli investimenti strategici, sostenuto fortemente anche dall'Italia. La flessibilità necessaria sull'utilizzo dei fondi esistenti, PNRR compreso, si accompagna all'altro grande tema oggi sul tavolo, decisivo per l'Italia, che è la revisione del Patto di stabilità e crescita. C'è ancora del lavoro da fare per finalizzare la revisione, ma riteniamo fondamentale arrivare entro il 2023 a nuove regole per dotarsi di principi credibili, realistici e coerenti con la situazione *post*-Covid. Stabilità e crescita meritano finalmente un equilibrio effettivo. Abbiamo avuto un Patto di stabilità e crescita che negli anni passati era molto più attento al tema della stabilità; oggi abbiamo bisogno di attenzione al tema della crescita questa deve essere la nostra priorità. Le vecchie regole sarebbero oggi assolutamente irrealistiche e quelle quelle nuove devono invece sostenere con efficacia i considerevoli investimenti pubblici necessari in questi anni in tutti i settori strategici, compresi l'ambiente, la difesa, la digitalizzazione. Il tempo dell'austerità è finito e il percorso di riequilibrio dei bilanci pubblici degli Stati maggiormente indebitati non dovrà sacrificare la dimensione dello sviluppo economico, non solo per evitare di colpire ulteriormente famiglie e imprese, ma perché la crescita economica stabile e duratura è anche l'unica vera garanzia di sostenibilità del debito pubblico. Il Consiglio europeo affronterà nuovamente anche il tema della sicurezza energetica, con l'obiettivo principale di valutare l'efficacia delle azioni intraprese finora e di verificare lo stato di preparazione in vista del prossimo inverno. L'Italia, fin dal principio, ha sostenuto l'importanza di una risposta a ventisette, con strumenti e obiettivi comuni tesi a rafforzare il sistema energetico nel suo complesso; la diversificazione delle fonti, in particolare del gas naturale; la lotta contro la speculazione e le disfunzioni del mercato del gas, volta a ripristinare un livello di prezzi ragionevoli per famiglie e aziende europee; la riduzione della domanda energetica; l'accelerazione dello sviluppo e della diffusione delle rinnovabili; il rapido riempimento degli impianti di stoccaggio. La decisione dell'Unione europea, fortemente "lavorata" e perseguita dall'Italia, di fissare un tetto massimo al prezzo del gas ha interrotto i fenomeni speculativi ai quali avevamo assistito nei mesi scorsi, con un enorme beneficio per le famiglie e le imprese italiane ed europee. È in gran parte un merito dell'Italia

Nelle conclusioni del Consiglio europeo vi sarà, infine, un riferimento allo sforzo europeo per le popolazioni colpite in Turchia e Siria dal recente terremoto. L'Italia, come sapete, ha prontamente risposto con l'invio di squadre di soccorso della Protezione civile e dei Vigili del fuoco, di beni e di contributi finanziari. Ha partecipato, ieri, alla Conferenza dei donatori, in uno spirito di vicinanza e solidarietà, nei confronti sia del popolo turco che di quello siriano. Continueremo, anche qui, a fare il nostro lavoro. In conclusione, colleghi, la voce dell'Italia è e sarà sempre più una voce forte in Europa. È questo il mandato che abbiamo ricevuto dai cittadini ed è questo il mandato che intendiamo portare avanti nei prossimi cinque anni. L'Italia vuole tornare a essere una nazione protagonista nel contesto europeo, anche per fare la sua parte nel rafforzare e migliorare la casa comune europea. Questo è quanto intendo rappresentare al Consiglio europeo, ovviamente col sostegno del Parlamento italiano e con il mandato che ci darete oggi. *(Applausi)*.

alla vigilia del Consiglio europeo voglio esprimere il ringraziamento per la lucida attenzione con la quale il Governo e il Presidente del Consiglio stanno trattando gli argomenti in agenda. è un ringraziamento non scontato, non di appartenenza, perché in casa nostra, come si sa, non esistono *yes men*, ma si misurano le azioni e si premiano i meriti, l'impegno, la coerenza e non la propaganda fine a se stessa. Nel solco della coerenza, la posizione di Fratelli d'Italia sul conflitto ucraino rimane la stessa che predicavamo dai banchi dell'opposizione. Eppure sarebbe stato facile assumere una posizione diversa da quella del Governo che ci ha preceduto; sarebbe stato magari empatico cavalcare l'onda di coloro (e ce ne sono anche in questa Assemblea) che esprimevano timidi rimbrotti nei confronti del presidente Putin o di coloro che con costanza disprezzano lo scudo della NATO. Ma noi non siamo timidi e le cose le diciamo con chiarezza. La visita del Presidente del Consiglio di alcune settimane fa ha suggellato la ferma posizione dell'Italia a fianco del popolo ucraino, il sostegno multidimensionale a quel Paese, l'impegno nel processo di ricostruzione, volto ad evitare la strumentalizzazione della sicurezza alimentare, perseguendo, pari tempo, le iniziative volte a far cessare le ostilità, con un traguardo che deve avere sempre come bandiera il sacrosanto principio di autodeterminazione dei popoli. In tal senso, guardo con sospetto qualsiasi iniziativa politica alternativa a quella dell'Occidente e ancor più la legittimazione del ruolo del capo del Cremlino da parte di Xi Jinping, perché il timore è quello che ci si liberi dall'abbraccio mortale della madre Russia e si venga soffocati dai tentacoli della madre "Ru-xia". L'Italia, il nostro Paese, in questo contesto giocherà un ruolo fondamentale, perché oggi è in grado di esprimere una propria posizione, è in grado di difendere la sovranità italiana senza mai far venir meno la collaborazione con le altre Nazioni d'Europa. È questo il cambio di marcia del Governo Meloni: essere autorevoli e non autoritari, agire con sussiego e non con tracotanza, ma soprattutto avere ridato dignità al pensiero della Nazione che finalmente si spoglia del ruolo ancillare al quale per diversi aspetti e su diversi piani era stata relegata. Agire nell'interesse della Nazione non significa essere contrari all'Unione, significa invece non abdicare, in forza degli interessi diversi e confliggenti, a difendere i princìpi sacrosanti della propria identità e della propria cultura, che peraltro sono quelli riportati nella Carta del Trattato istitutivo, che si rispetta e non si interpreta a seconda dei momenti e delle opportunità. Per questo siamo convinti che il nostro Presidente del Consiglio saprà imprimere al dibattito e all'agenda quella giusta direzione che per anni era stata declinata a vantaggio sicuramente delle banche, delle multinazionali, delle organizzazioni non governative, della corrente del pensiero del *mainstream*. Pretendere la revisione della legge di stabilità e delle regole dei cosiddetti aiuti di Stato non è cavalcare l'onda di una protesta antieuropeista, tutt'altro. Chi azzarda un simile paragone non ha compreso i temi del dibattito o è in ostinata malafede, perché è proprio dalla volontà di adeguare le regole all'impegno massiccio della cosiddetta ricostruzione *post* pandemia che si misurerà la volontà di lavorare per un'Europa unita e non per singole aggregazioni di potere. Dobbiamo liberarci dalle farisaiche dichiarazioni di facciata e pretendere che in concreto, di fronte a un cambio epocale, non vi sia chi per interessi di bottega si opponga al *price cap* o a salvaguardare il In questo contesto, appare sicuramente strano relegare il tema dei migranti tra le varie ed eventuali attuali e non come un tema all'ordine del giorno, manifestando così, senza ogni ragionevole dubbio, la distanza dell'Europa dal problema e l'apollinea estraneità alla questione di chi ha fissato l'ordine dei lavori. Per noi, invece, l'emergenza migranti è in cima alla lista dell'agenda, perché nei fatti e non nella propaganda elettorale vogliamo evitare il ripetersi di tragedie come quella di Cutro, guardando la luna e non la punta del dito come qualcuno scriveva nei giornali oggi, perché non può esserci un'Europa che condanna l'Italia ad essere l'unico presidio per i popoli migranti e non censura l'atteggiamento dei Paesi dell'Europa che negano l'approdo sulle loro coste o vogliono farci credere che la rotta balcanica arrivi in elicottero nel mio amato Friuli-Venezia Giulia. Questa non è l'Europa di solidarietà che noi vogliamo e siamo certi che il presidente Meloni saprà imprimere questo cambio di passo, perché rispetto al passato c'è un fattore che più di ogni altro qualifica l'operato di questo Governo ed è quello del Presidente del Consiglio. Noi non siamo portatori di interessi, non agiamo in nome e per conto delle organizzazioni di profitto, vogliamo dare legittimità al flusso dei migranti e sul rispetto delle regole avulse dal profitto siamo in grado di dare la nostra autorevole testimonianza. *(Applausi)*.

Ci siamo visti in occasione della sua prima venuta a dicembre e abbiamo parlato del tema migrazione, che è particolarmente centrale. Mi permetto di dirlo di dirlo a lei, ai tanti colleghi e ai cittadini italiani: i popoli, gli esseri umani migrano da oltre due milioni di anni per vari motivi, tra cui anche quelli economici. *(Applausi)*. Pertanto, il tema della migrazione non è una novità,

e, essendo un lembo d'Africa insicuro, continua a essere una spina nel fianco per l'Italia e per il confine meridionale dell'Europa.

un rapporto equilibrato con gli amici francesi, dopo che ha parlato di questo negli ultimi quattro anni? Il problema delle migrazioni è serio e va affrontato in maniera adeguata. Abbiamo visto che

L'altra grande questione legata alle migrazioni è quella economica. Come pensiamo di affrontarla? Lei ha fatto un cenno nella sua relazione. Affrontiamola in maniera unitaria e solidale, perché non è solo bloccando - non so come - i flussi primari che si risolvono i problemi dei flussi secondari: mi sembra una battuta alla Catalano e mi dispiace essere così diretto.

Lei ha detto: «Attaccate me, non attaccate l'Italia». Noi siamo sempre e assolutamente al fianco dei cittadini italiani, non abbiamo nessuna intenzione di attaccare l'Italia e, se attacchiamo lei e il suo Governo, lo facciamo su basi oggettive. Ha visto i flussi migratori degli ultimi mesi verso l'Italia, dopo che lei ha fatto proclami, ha attaccato le ONG, ha parlato di blocchi navali e poi fortunatamente ha fatto marcia indietro. I blocchi I blocchi navali, o comunque i muri galleggianti, non possiamo metterli. È un problema legato al confine meridionale, che va difeso in maniera adeguata. Altra cosa è il problema dei confini balcanici.

Era un viaggio ovviamente simbolico, per dire buon lavoro a lei e a tutti gli italiani. In realtà lei ci ha preso molto sul serio, perché - spero di non dimenticare nulla - in pochi mesi è andata in Albania, in Algeria, in Egitto, negli Emirati Arabi Uniti, in India, in Iraq, in Libia e in Ucraina, oltre ovviamente agli appuntamenti internazionali a Bruxelles e con gli altri *partner* europei in Polonia, Germania e Svezia. Questi suoi viaggi, però, non sono stati semplicemente delle strette di mano, delle fotografie, dei motivi per fare notizia. Lei è tornata sempre con accordi commerciali, con accordi diplomatici e con accordi politici che hanno rafforzato il nostro Paese, ma soprattutto ha lanciato un messaggio: l'Italia c'è, l'Italia è tornata protagonista *(Applausi)*, l'Italia, soprattutto in alcune zone di mondo, torna a dire la sua come *partner* affidabile, in una cornice internazionale condivisa. Oggi all'ordine del giorno del Consiglio europeo troviamo ovviamente l'Ucraina

Questo significa per noi dare seguito a una affidabilità internazionale nei confronti della NATO, dell'Unione europea e di tutti gli accordi internazionali di cui facciamo parte. Non è stato sempre così, Presidente. L'Italia, grazie a questo Governo, è tornata nuovamente credibile sugli scenari internazionali; oggi siamo visti sicuramente in maniera differente e possiamo lavorare sia sul piano della difesa militare dell'Ucraina, ma anche per costruire un'ipotesi di pace. Per quello che riguarda la transizione verde, come lei ben sa (visto che è il nostro Presidente), noi facciamo parte del Partito dei conservatori europei. Più che un partito è una famiglia, una filosofia, uno stile di vita, una concezione della vita e del mondo. Noi siamo conservatori perché vogliamo conservare i valori fondamentali, innovandoli e proiettandoli nel futuro. Figuriamoci se non vogliamo conservare l'ambiente, se non vogliamo conservare il mondo in cui viviamo o se ci possiamo arrendere a un'ideologia che consuma e sfrutta territorio, suolo, aria e acqua. La nostra difesa dell'ambiente significa tutelare le nostre comunità, la nostra storia, la nostra identità. Ma tutto questo cosa c'entra con provvedimenti che, in nome di un'ideologia verde, rischiano di mettere in crisi settori strategici fondamentali della nostra industria, come quella automobilistica italiana ed europea? Grazie al nostro Governo e insieme ad altri Governi abbiamo fermato questa

mentre noi continuiamo a farci del male, imponendoci dei limiti incredibili, perché ovviamente dovremo rivalutare e rimodellare qualunque altra cosa, altri Stati, quelli più inquinanti, questi problemi non se li pongono proprio. È un modo, ancora una volta, per mettere l'Italia e l'Europa in difficoltà. Questo è quello che ci aspettiamo - come lei ci ha detto dal suo intervento al Consiglio europeo. Infine c'è il tema dell'immigrazione. Ringrazio il collega Lorefice, che ci ha ricordato che storicamente le migrazioni esistono da tempo, da decenni, anzi da secoli e da millenni. Proprio per questo - pensi - ho trovato una poesia. Addirittura centocinquanta anni fa il buon Edmondo De Amicis scriveva: «Ammonticchiati là come giumenti / sulla gelida prua morsa dai venti, / migrano a terre inospiti e lontane; / laceri e macilenti, / varcano i mari per cercar del pane. / Traditi» - pensi un po' - «da un mercante menzognero, carne da cimitero, / vanno a campar d'angoscia in lidi ignoti». Questa poesia ci ricorda appunto che i fenomeni delle migrazioni non nascono oggi. C'è stato qualcuno, qualche personaggio sinistro in tutti i sensi, che addirittura ha pensato bene di accollare la tragedia di Cutro

Noi ambiamo a pensare che questa poesia possa diventare storia, nel momento in cui qualcuno se ne prenderà carico, perché o l'Unione europea su questo farà la sua parte, oppure questa poesia sarà sempre, purtroppo, terribilmente attuale ai vari scenari dipinti, forse un po' di storia fa bene: la Libia ha avuto il suo momento critico, perché non solo un Governo, ma un intero Parlamento e un intero sistema politico diede il via libera libera a una guerra a quello che veniva ritenuto un grande e pericoloso dittatore. Noi oggi, Presidente, le diamo un ulteriore mandato. Oggi è il primo giorno di primavera e in in Italia, oltre alla primavera atmosferica, si respira anche una primavera politica: c'è un risveglio di progettualità, di riforme e un cambio di passo. Noi le auguriamo di poter portare questo senso di primavera un po' anche nella grigia e triste Bruxelles, ricordando all'Unione europea il motivo per cui è nata, cioè dare vita ad una sfida globale, trovando le soluzioni del caso. Grazie a questo, anche la voce italiana, che lei ci assicura essere sempre più forte,

i numeri sono impietosi e ci dicono che gli sbarchi, da quando governa la destra, sono quadruplicati. Ci avete accusato per anni di favorire un'invasione e avete gridato alla sostituzione etnica: non era invasione allora e non lo è nemmeno oggi. Smettiamola con la propaganda. Nessuno è in pericolo, tantomeno le nostre radici cristiane, a cui - mi creda - tengo anch'io. *(Applausi)*. Sono invece del tutto inadeguate le modalità con cui si tenta di affrontare un'emergenza immigratoria che avrebbe bisogno di ben altri visioni e strumenti per farvi fronte in modo efficace. Si dovrebbe in primo luogo evitare che decine e decine di profughi, in fuga da guerre, terremoti e dittature, arrivino a cento metri dalle nostre coste e trovino la morte, invece di trovare un nuovo inizio. Chi ha agitato lo spauracchio dell'invasione per cercare consenso, fomenta la paura dell'opinione pubblica e inquina - come stiamo già vedendo - con una propaganda distorta. Siete al Governo e spetta innanzitutto a voi il compito di governare i flussi migratori, che non possono rispondere a visioni politiche anacronistiche e discriminatorie. Siamo anche noi dell'avviso che l'Europa non può più, in questo contesto, comportarsi come ha fatto finora. Anche l'Europa ha grandissime responsabilità ed è chiamata a svolgere quel ruolo di guida essenziale quando parliamo di sicurezza, non delle frontiere italiane, ma di quelle, appunto, dell'Unione europea. Oggi bisogna sciogliere il nodo Tunisia, che sappiamo quanto sia complesso e non bastano un paio di motovedette. C'è da dire però, Presidente, che la destra guarda all'Europa solo quando deve chiedere, come accade adesso. Ricordiamoci la questione dei ricollocamenti, mai attuati a causa della contrarietà dei vostri vostri alleati europei, i Paesi di Visegrad, che sul tema dell'immigrazione hanno saputo bene scaricare la responsabilità su altri, lavandosene le mani, e contestualmente erigere inutili e antistorici muri che offendono la storia degli europei e voi dietro a loro. Dall'Europa si si deve pretendere giustamente che si assuma le proprie responsabilità, ma l'Italia lo potrà fare con assoluta legittimità solo se non romperà l'unità della Comunità dei ventisette e terrà salde le alleanze strategiche di Roma. Il Governo potrà chiedere se avrà dimostrato di essere coerente con una visione che fa dell'accoglienza e dell'integrazione non due vessilli su cui sparare, com'è successo per anni, ma rimuovendo normative assurde, come la legge Bossi-Fini, che gli stessi autori considerano superata. Cosa aspettate a cambiarla? Lo stesso sottosegretario Mantovano ha dovuto ammettere che quella legge non ci serve. Con quale credibilità, Presidente, si presenterà al Consiglio europeo a rappresentare il Paese, avendo sinora prodotto solo uno - sbagliatissimo - decreto, che offende che offende l'intelligenza di noi europei? Certo, anche noi siamo per combattere gli scafisti, che sono però un problema conseguente; noi dobbiamo andare alla causa. Sull'immigrazione occorre cambiare rotta o il Paese si ritroverà dentro una crisi umanitaria senza precedenti. Presidente Meloni, le persone in mare vanno salvate sempre e senza pensarci nemmeno un secondo. Ora però l'Italia si presenta in Europa avendo sulla coscienza due tragedie che potevano essere evitate; quella immane di Cutro e quella altrettanto grave del barcone che, fuori dalla Libia, ma in acque internazionali, si è ribaltato mentre sopraggiungevano nostri mercantili, ai quali

che l'Europa ci ascolti. Ve lo chiedo anch'io: perché quelle persone sono morte quando potevano essere salvate? Cosa non ha funzionato quella notte davanti alla spiaggia di Cutro? Dove è mancata la catena di comando? Ancora nulla sappiamo, ma, come dice Pasolini, tutti sappiamo, ma non abbiamo ancora le prove. Comunque la verità verrà a galla. Servono corridoi umanitari; serve, quello sì, un nuovo decreto flussi che riveda le quote di immigrati regolari che possono entrare nel nostro Paese perché di fronte a perseguitati politici, a famiglie che fuggono da zone di guerra, da terremoti o da situazioni insostenibili, noi abbiamo il compito di dare accoglienza e di aiutare queste persone - uomini, come noi, ma più sfortunati di noi - a trovare una sistemazione dignitosa, ben sapendo che solo uno su dieci si fermerà nel nostro Paese. Sono infatti persone in fuga, alla ricerca dei propri cari, che vivono per lo più in Germania, in Francia e nel Nord Europa. Questo è l'unico modo per andare in Europa a testa alta per chiedere aiuto. Se invece continuerete sulla strada della retorica e della propaganda, le cose peggioreranno sempre di più; cambiate rotta. Voglio infine ricordare a noi tutti c'è un'altra emergenza migranti, oltre a quella che sta flagellando il mar Mediterraneo e si trova a Nord-Est della penisola; è la rotta balcanica che, anno dopo anno, è diventata una delle porte di accesso più battute per entrare in Europa e, in particolare, in Italia. I numeri si impennano mese dopo mese; afgani, pakistani, turchi - curdi in particolare - ma anche somali, marocchini, bengalesi. In questi primi mesi dell'anno sono entrati nella mia Regione, il Friuli-Venezia Giulia, quasi 2.400 migranti dal Carso triestino, dalle colline goriziane, dalla montagna tarvisiana e dalle valli del Natisone. Lo scorso anno erano stati, nello stesso periodo, meno di 900; ma cosa facciamo? Alziamo un bel muro tra noi e la Repubblica di Slovenia? Lo proponeva la giunta del presidente Fedriga che oggi vuole fermare il flusso via terra con 65 fototrappole. Avete sentito bene: 65, piazzate in decine e decine di chilometri di boschi. Ancora propaganda elettorale. Ecco, sforziamoci di essere seri e pragmatici, diamo risposte all'altezza di tali fenomeni. Fino al giorno delle elezioni proponevate un blocco navale, che sapevate impossibile; ora avete l'onere di creare un consenso europeo sulle politiche di gestione dei flussi migratori che coinvolga il Mediterraneo e i Balcani.

Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare moltissimo il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per aver voluto fornire questa informativa alle Camere, e quindi agli italiani, prima di recarsi al Consiglio europeo: un atto di attenzione e di condivisione, che sottolinea l'importanza e la centralità che il Governo intende dare al Parlamento e al suo ruolo. un passaggio preliminare tanto più importante, perché importanti e rilevanti sono le questioni che l'Italia si appresta a portare in questo Consiglio europeo. È un'Italia che vola a Bruxelles, come è volata in tanti luoghi del mondo, in questi primi quattro mesi di legislatura, con idee chiare, con proposte concrete, pronta a dare il proprio contributo fattivo alla risoluzione delle grandi criticità che attanagliano l'Europa e che ci riguardano tutti. criticità vanno affrontate e risolte nel contesto europeo, ma è bene sottolineare che sono criticità che interessano e investono, in primo luogo, come nel caso del dramma dell'immigrazione, principalmente proprio l'Italia. Mi auguro che questo grande sforzo del Governo italiano per avere risposte positive dall'Europa possa essere accompagnato da un'attenzione corale e non pregiudizievole anche dalle forze politiche che rappresentano l'opposizione, perché in gioco ci sono tematiche estremamente rilevanti e destinate a incidere sul futuro della nostra Nazione e degli italiani di oggi e di domani. Andiamo in questo Consiglio europeo con delle proposte concrete che portiamo all'attenzione dell'Europa: già questa è una rilevante novità. Spesso l'Italia non aveva una propria voce, spesso rimaneva muta, spettatrice supina di decisioni non propriamente condivisibili che non andavano esattamente incontro al nostro interesse nazionale. Non doveva essere così e oggi, fortunatamente, non è più così. Oggi c'è un Governo che non solo porterà a quel tavolo le nostre proposte, ma che ha lavorato affinché si possa raggiungere una sintesi ampia fra gli Stati dell'Unione europea, affinché il punto di vista italiano possa avere l'attenzione che merita e possibilmente essere fatto proprio dall'Europa. Porteremo delle soluzioni concrete sul tema dell'immigrazione, perché è di tutta evidenza che serve una gestione finalmente europea dei flussi migratori, nel controllo delle frontiere, nella cooperazione sui rimpatri, nella lotta all'immigrazione clandestina, colpendo con durezza gli scafisti e tutti coloro che guadagnano e lucrano sul traffico di esseri umani, provocando lutti e tragedie come l'ultima di Cutro. Ribadiremo la nostra linea sull'Ucraina affinché, mai come oggi, l'Europa possa continuare ad essere ferma e vigile nel sostegno ad una Nazione invasa. C'è il tema della transizione verde e digitale, che va rimodulata, mediante un percorso che sia realmente sostenibile sul piano economico e sociale. Daremo le nostre idee per una transizione ecologica rispettosa del sistema produttivo, tenendo conto dell'esigenza dell'Italia e dell'Europa di realizzare l'autonomia strategica europea, limitando le dipendenze dalle materie prime e dalle tecnologie di Paesi extraeuropei, ma va garantita adeguata considerazione della specificità degli Stati membri. Con la direttiva sull'efficienza energetica nell'edilizia, facente parte delle misure da adottare nell'ambito Fit for 55, il Consiglio e il Parlamento europeo stanno discutendo l'introduzione di *standard* minimi di prestazione energetica degli edifici irrealistici per l'Italia e per questo il Governo interverrà per rivedere la portata di tale direttiva. Faremo ascoltare la nostra voce sui temi economici, sulla riforma della *governance* europea, sul nuovo patto di stabilità, che deve garantire la flessibilità dei fondi europei e su questo andrà trovato un accordo. Vogliamo sostenere il negoziato sulla riforma della *governance* e auspichiamo che siano valorizzate le indicazioni contenute negli atti di indirizzo approvati dai due rami del Parlamento italiano. Devo dire che la Commissione bilancio ha svolto un lavoro piuttosto complesso sul tema e deve essere adottato un approccio che tenga conto del ricorso all'uso flessibile dei fondi europei, adeguando gli obiettivi della politica di coesione al sostegno di tutti i fattori abilitanti la crescita economica e la competitività del nostro Paese e dell'Europa, a partire dal nostro tessuto industriale. Concludo l'intervento, Presidente, dicendo che siamo assolutamente con il presidente Meloni nel ritenere che vi debbano essere svolte di grande rilievo. Siamo fiduciosi che il lavoro complesso che si sta portando avanti possa portare a importanti risultati per la nostra Nazione. (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, onorevoli Ministri, colleghi senatori, presidente Meloni, le sue comunicazioni in previsione del Consiglio europeo dei prossimi 23 e 24 marzo rispecchiano appieno la sua cifra umana, il suo carattere politico e rispecchiano anche le aspettative che milioni di italiani hanno riposto L'Italia è orgogliosa di lei perché, con la preparazione e la determinazione che la contraddistinguono, è già riuscita - le do una notizia *ictu oculi* - a riportare l'Italia al ruolo di protagonista dell'iniziativa politica europea, che ancor più con la guerra, con la crisi energetica e oggi bancaria, si dovrà distinguere per la velocità delle decisioni e per la realizzazione di una visione non burocraticistica, ma condivisa con i popoli europei che sono stati spesso delusi dalle scelte dei vertici dell'Unione, più propensi ad occuparsi della farina di grillo piuttosto che delle vere emergenze. riferisco, appunto, all'immigrazione, alla realizzazione di una politica estera e di difesa comune forte, capace di garantire la sicurezza del Continente e la promozione di un'economia di sviluppo sana, della crescita, come da lei citata, dove l'anima e le aspettative dei cittadini suppliscano piuttosto al mero e freddo calcolo finanziario. La credibilità che, nel breve tempo, dall'inizio del suo Governo, è riuscita a rivendicare a livello comunitario e internazionale, che ha allarmato le opposizioni in cerca di un *casus belli*, ha fatto in modo che, per la prima volta, l'Europa abbia realmente capito, dopo il tragico naufragio di Cutro, che i confini dell'Italia sono i confini dell'Europa intera, che il fenomeno dell'immigrazione di massa è un'ondata che, come dice Panebianco oggi, rimetterà in discussione il concetto stesso di Nazioni e di Unione europea. Questa consapevolezza non solo ha posto al centro del tavolo il problema dell'immigrazione massiccia verso il nostro Paese, ma ha anche consentito, grazie al suo intervento, l'erogazione straordinaria di oltre 500 milioni di euro, confermati proprio in queste ore dalla presidente von der Leyen, volti a tamponare il disagio geopolitico proprio dell'Italia e l'enorme fardello che siamo costretti, ormai da troppi anni, a sopportare, non senza colpevole responsabilità dell'Occidente. Gheddafi lo aveva detto: la Libia è l'ultimo argine contro la transumanza dell'Africa in Europa. Nel suo intervento, la presidente Meloni ha illustrato con chiarezza la linea che dovrà essere intrapresa su questo fronte: supportare i Paesi di partenza - penso in particolare oggi alla Tunisia, che è sull'orlo di una crisi che potrebbe generare una nuova ondata di migranti - ma al contempo pretendere da quegli stessi Paesi serietà e responsabilità. Non sono più tollerabili porti franchi ed è prioritaria la lotta agli scafisti e ai loro mandanti. Ciò anche alla luce delle ultime inquietanti notizie - tutte da accertare - secondo cui addirittura Ministri di alcuni di questi Paesi che noi aiutiamo sarebbero gestori stessi dei trafficanti. Fatti come questi - se confermati, appunto - sono inaccettabili e ingiustificabili e alimentano quel senso di sfiducia dei cittadini rispetto al fenomeno migratorio che l'Europa deve combattere. Ecco come l'Unione può dimostrare di esistere e di non essere solo un centro di compensazione di interessi; organizzare finalmente una gestione europea dei flussi migratori, dal controllo delle frontiere alla formazione dei migranti, alla cooperazione sui rimpatri, alla lotta agli scafisti e all'integrazione. Siamo soddisfatti del tempestivo decreto-legge che il Governo da lei guidato, Presidente, ha posto in essere nell'importante e simbolico Consiglio dei ministri tenutosi a Cutro all'indomani del naufragio, che non è dovuto, colleghi, al Governo, con il quale è emersa una verità taciuta in tutta la polemica strumentale seguita e da me già messa in evidenza prima di chiunque altro in quest'Aula: i responsabili di questo martirio umano sono i trafficanti di morte e non, come dice chi fa sciacallaggio, i Governi, in particolar modo il nostro, che, a differenza di altri Stati membri, come la Grecia o la Spagna, accolgono incessantemente e senza alcun respingimento i disperati che arrivano o transitano sul nostro territorio. Su questi temi che investono l'interesse dell'Italia maggioranza e opposizione dovrebbero trovarsi sempre sullo stesso fronte. Lei lo ha chiesto e gli italiani lo sperano, Presidente. È ancora fondamentale rilevare l'attenzione dimostrata nella riapertura dei flussi e nel riconoscimento di un'immigrazione necessaria necessaria al sostentamento del nostro Paese, ma altrettanto fondamentale è la formazione che dobbiamo promuovere prima che costoro partano per venire a lavorare in Italia. Sulla situazione in Ucraina è umano e naturale, per la salvaguardia dei nostri principi democratici, rivendicare il nostro sostegno al Paese aggredito, fornendogli tutti gli strumenti utili alla difesa necessaria, necessaria, ribadendo che ogni possibile soluzione di pace passa dall'integrità territoriale dell'Ucraina. Al contempo, però, auspichiamo che il nostro Paese assuma ancora una volta quel ruolo di ponte tra le nazioni per la realizzazione di una pace giusta e duratura, che promuova il dialogo esaltando il nostro tradizionale ruolo di esportatori di pace. Avviandomi alla conclusione, signor Presidente del Consiglio, la sua sensibilità verso le fasce più deboli dei cittadini è nota e anche la sua abnegazione nel raggiungere successi politici giusti e insperati; pertanto, nel Consiglio europeo, oltre a reiterare la necessità di una maggiore flessibilità dei fondi di stabilità, la prego di farsi carico dell'urlo strozzato di migliaia di cittadini europei, ma soprattutto italiani, per la miope - me lo si lasci dire - politica della presidente della BCE Lagarde, che è notizia di oggi stia correndo ai ripari dei danni da lei stessa arrecati. In conclusione, serve veramente un suo autorevole e personale *whatever it takes* per svegliare le coscienze

i cambiamenti climatici sono la più grande sfida che siamo chiamati ad affrontare nell'immediato e nei prossimi anni. Purtroppo le conseguenze sono già sotto gli occhi di tutti: cito solo il caso della forte siccità che sta colpendo il Veneto, il Lago di Garda, l'Adige, il Po, le Regioni del Nord Italia. Siamo molto preoccupati, sappiamo che la siccità non aspetta i comodi di nessuno, tantomeno i tempi del suo Governo. Sono passati infatti cinque mesi dall'inizio della legislatura e non è un mistero per nessuno il fatto che in cima alla vostra agenda non avete messo tutte quelle azioni di contrasto al cambiamento climatico che sta aumentando la temperatura globale e alterando l'ambiente in cui viviamo, l'economia, le comunità e non ultima la nostra salute. Mi preme dirlo subito e ripeterlo ancora perché urge un cambio di rotta: non c'è più tempo da perdere. Certo, questa sfida impone scelte coraggiose, competenti e lungimiranti, come ha detto anche lei, signora Presidente del Consiglio, ma non siamo soli ad affrontarla. L'Unione europea sta promuovendo la transizione verso un continente a basse emissioni di carbonio, facilitando investimenti pubblici e privati nell'energia pulita. Questo indirizzo si regge sul principio che un settore energetico più pulito sarà catalizzatore di crescita e occupazione allo stesso tempo sarà più sostenibile, più sicuro e capace di alleggerire le bollette dei cittadini. Sembra ed è un obiettivo raggiungibile, invece non lo è perché questo Governo, chiamato a rappresentare gli interessi del nostro Paese in Europa, sta andando in direzione totalmente opposta. Purtroppo ho solo tre minuti e non posso elencarlo, ma l'ultimo esempio è dato dal fantomatico progetto di creare l'*hub* di approvvigionamento energetico d'Europa, continuando ancora a puntare sui fossili. Le decisioni in ambito energetico che questo Governo sta assumendo sono preoccupanti e inoltre sono semplicemente miopi. Di fatto state scaricando sulle future generazioni le conseguenze di queste scelte, *in primis* quella di non voler diminuire i sussidi nei confronti dei combustibili fossili, responsabili dell'aumento dei livelli di produzione dell'inquinamento. Signora Presidente del Consiglio, le chiedo di far pubblicare finalmente il catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e di quelli favorevoli; da circa un anno, infatti, il Ministero dell'ambiente lo tiene chiuso in un cassetto, nonostante la pubblicazione sia obbligatoria per legge. Il catalogo rappresenta la fotografia di come l'Italia abbia dirottato i fondi in materia ambientale e di come siano state promosse misure di *green economy.* Questa mancata pubblicazione sta mettendo l'Italia anche in una posizione di svantaggio in sede europea, quando bisognerà lavorare su questo genere di informazioni. Chiediamo infine che il Governo riferisca costantemente in Parlamento sullo stato di avanzamento della stesura del Piano nazionale integrato energia e clima, visto che entro giugno andrà presentato alla Commissione europea, affinché possa essere approvato dall'Unione europea con eventuali modifiche e infine approvato entro la fine del una questione importante, perché avrà ripercussioni sulla vita di tutti i cittadini. Signor Presidente, concludo dicendo che abbiamo il diritto di apprendere come questo Governo intenda raggiungere il taglio del 55 per cento delle emissioni di CO₂ entro il 2030, visto il costante rafforzamento della sua dipendenza da fonti

Signor Presidente, signora presidente Meloni, noi tifiamo per il suo successo in Europa, perché il suo è il successo del nostro Paese; lei non rappresenta le mie idee, ma rappresenta il Paese, quindi se lei riesce in Europa vuol dire che è riuscita l'Italia. Mi fanno piacere le sue parole secondo cui non si fa sciacallaggio politico, ma si hanno idee diverse. È così lontana la Giorgia Meloni che nel 2015 chiedeva che l'allora *premier* Matteo Renzi venisse indagato per strage colposa nel Mediterraneo, dopo il naufragio di una nave. *(Applausi)*. Siamo cresciuti tutti, siamo invecchiati tutti, quindi oggi ci preme portare a casa dei risultati. Chi parlerà dopo di me farà un discorso molto più ampio; a me interessa quello che lei ha detto sulla transizione ecologica,

azioni concrete. A chi pensa che la transizione ecologica debba essere sempre fatta senza se e senza ma, dico però che farla vuol dire fare delle scelte. noi siamo molto forti sull'energia rinnovabile dell'idroelettrico (siamo *leader* in Europa), ma lo siamo meno sulla produzione di pannelli solari. Allora, l'Europa si deve mettere in testa di fare una filiera industriale sulla transizione ecologica, altrimenti finiamo per passare dalla dipendenza dal gas russo alla dipendenza dalle terre rare cinesi. A chi pensa di essere ecologista più di noi, che andare verso la transizione ecologica vuol dire fare delle scelte, ad esempio aprire nuove miniere in Italia per l'estrazione di quelle terre rare che servono alla costruzione dei pannelli fotovoltaici. Perché dipendere dalla Cina, quando nel nostro Paese abbiamo quel materiale?

agricola e a quelle società che in questi anni hanno fatto del riciclo delle materie prime e seconde la nostra bandiera in Europa. Parliamo sempre male della nostra possibilità di raccolta rifiuti, ma in realtà siamo *leader* europei per la raccolta e il riciclo delle materie prime e seconde: abbiamo già raggiunto gli obiettivi del 2025 e del 2030. In Europa però, signora Presidente, dobbiamo fare una battaglia: a breve arriverà un regolamento

se sia felice dei Primi ministri spagnoli e francesi (probabilmente avrà fatto campagna elettorale per i loro antagonisti), ma oggi rappresenta il nostro Paese e Francia e Spagna hanno gli stessi nostri obiettivi, ossia indurre l'Unione europea a rivisitare completamente quel regolamento che, se venisse che, se venisse applicato così com'è stato scritto, sarebbe una tragedia per le nostre aziende agricole, per il nostro *export* (quest'anno abbiamo esportato per 52 miliardi) e soprattutto per chi in questi anni ha una battaglia di civiltà, facendoci raggiungere quell'economia circolare di cui - lo dico a Timmermans - tutti parlano, ma pochi evidentemente applicano e in cui l'Italia è molto più *leader* di altri Paesi, quindi non abbiamo bisogno di lezioni da nessuno.

il Gruppo Forza Italia appartiene al Partito popolare europeo ed è quindi portatore di una istanza europeista convinta. Tuttavia, ogni tanto, quando vediamo delle decisioni del Parlamento europeo, della Commissione europea e delle varie istituzioni, ci sorge qualche dubbio, non sull'europeismo, che non viene meno e che peraltro è antico, anche con percorsi vari, ma sul modo di decidere dell'Europa,

a volte, assisto trasecolato ad alcuni processi decisionali dell'Unione europea tali per cui sembra che si facciano le cose che vanno evitate e non si facciano quelle che si dovrebbero fare.

quella ipotesi di risoluzione. Lo stesso si potrebbe dire su altre vicende, ad esempio quelle riguardanti l'auto: è stato un successo del Governo italiano, che fa bene a rivendicare (se n'è occupata lei e se n'è occupato il ministro Pichetto Fratin), il rinvio della votazione sulla direttiva dell'auto, che prevede tempi e modalità improponibili e lesive. Sono proprio quelle scelte, come ha detto nel suo intervento, che rischiano di dare alla Cina e ad altri la potestà mondiale su alcune materie prime, ecco perché credo che

di rimettere le carte a posto. L'Europa deve rimettere le misure da evitare nella cartella delle misure da evitare e quelle da fare nella cartella giusta: difendere la casa, difendere il lavoro, difendere l'industria. Lei ha fatto un cenno alla concorrenza. Non è possibile che gli Stati Uniti, patria del capitalismo e dell'economia libera, stanzino centinaia di miliardi di dollari per le loro industrie e noi, invece, andiamo ancora a fare la guerra all'ultimo artigiano nel sospetto che ci siano gli aiuti di Stato. Lei lo ha detto, su questo bisogna essere più flessibili, ed è scritto nella risoluzione. Noi non vogliamo un'economia dirigista, non vogliamo un'economia dirigista, ma realista. Se oggi c'è un momento di crisi nel mondo, per le guerre e per l'energia, se gli americani aiutano le loro imprese e i cinesi fanno concorrenza sleale a tutto tondo, noi dobbiamo difendere l'Europa, le imprese e l'economia europee,

L'Europa deve far pagare le tasse a Google e ad Amazon, ai padroni del mondo che pagano praticamente zero tasse. Invece di prendersela con i bagnini, si occupino di Bezos e di quelli che stanno alterando la concorrenza e non pagano tasse. L'Europa ha in programma ma evidentemente il relativo foglio era andato nella cartellina sbagliata. Voglio anche dire al Governo che oggi leggo affermazioni di Gentiloni di Timmermans, che ci accusano di un errore ideologico in materia d'inquinamento: ma è proprio gente come Timmermans che pensa che il cambio delle automobili avvenga domani o che le case vadano ristrutturate dopodomani a spese degli italiani. ad essere affetti da un ecologismo ideologico, mentre noi vogliamo una tutela dell'ambiente reale, seria, possibile e praticabile, quindi è inutile che oggi Timmermans faccia la lezioncina

ci dicevano: sì, la Francia è arrabbiata, ma guardate quanto è bravo Macron. Ora abbiamo una Francia in rivolta e ingovernabile e l'Italia ha ottenuto in Europa il successo del prezzo del gas: è Macron che deve fare il maestro con noi o noi che possiamo dare qualche consiglio alla Francia?

Cina. Dobbiamo guardare anche alla storia. Il sostegno al popolo ucraino è totale, abbiamo votato e voteremo tutte le misure necessarie e abbiamo fatto e faremo la nostra parte, ma l'Europa un obiettivo di dialogo di pace se lo deve pur dare o vogliamo lasciare alla Turchia e alla Cina il ruolo di negoziatori del pianeta? Noi siamo l'Europa, dobbiamo sostenere i popoli aggrediti, ma indicare anche un percorso di pace all'umanità, perché serve ai nostri popoli e alla nostra economia. Sull'immigrazione ovviamente siamo totalmente d'accordo. Visto che dalla Libia,

quattro Gheddafi sono peggio ancora: questo è successo in Libia, con tutti i riflessi sui flussi incontrollati. La von der Leyen ha scritto una lettera - e ha fatto bene - frutto anche degli impegni e delle sollecitazioni rivolti dal Governo italiano e dalla presidente Meloni: Meloni: servono soldi e la difesa dei confini europei. Aggiungo, presidente Meloni, che ieri nel Consiglio dei ministri degli esteri il vice presidente del Consiglio Tajani ha sollecitato quell'intervento per la Tunisia. Noi dobbiamo vedere l'Europa e il Fondo monetario agire in Tunisia, perché, se la Tunisia affonda, i 200.000-300.000 tunisini pronti a fuggire vengono in Italia e poi al Fondo monetario ad altri non importa niente. Poi noi veniamo messi sotto accusa, se non accogliamo tutti? Ci

politico, oltre che rimettere le carte nelle cartelline giuste ed evitare che l'Europa faccia il contrario di quello che deve fare nell'interesse dei suoi popoli, perché o si affrontano

non solo venga rafforzata l'istituzione europea - oggi ne parla Panebianco sul «Corriere della sera» - ma che ci sia anche una maggioranza europea di centrodestra. questo le elezioni europee del 2024 sono importanti. Che si ricordi di difendere i nostri produttori, i nostri confini marittimi, le nostre case, il futuro dell'Europa e quindi anche dell'Italia.

Presidente Meloni, lei chiede collaborazione da parte dell'opposizione. L'opposizione collabora, a patto che però non si venga in Senato a prendere in giro gli italiani: lei dice che non stiamo spendendo un euro

Lei deve dirci con quali soldi reintegrerete il nostro arsenale militare. Presidente Meloni, lei viene qui a dirci che tutta l'Europa sta pagando il prezzo dell'aggressione russa, aggiungendo anche che tutti noi dobbiamo fare la nostra parte: questo potrebbe anche essere corretto,

Capita infatti - e lei lo sa benissimo - che la Germania si è fatta passare un piano di sostegno economico da 200 miliardi e la Francia uno di poco meno. Lei oggi, invece, si presenta qui con i numeri

Presidente Meloni, non so se palazzo Chigi può essere qualcosa di molto distante, ma fuori da qui c'è un carovita che è diventato insopportabile: si parla di 3.000 in più annui a famiglia, per non parlare poi della scellerata decisione della BCE di alzare i tassi. Si pensi che in questo momento si parla di una vera e propria tassa patrimoniale sulla casa, perché, se consideriamo l'aumento dei ratei e lo spalmiamo per tutta la durata del prestito, abbiamo una tassa patrimoniale per famiglia di 60.000 euro. *(Applausi)*. Questi sono i problemi ai quali lei si deve rivolgere. altro che operazione militare; qui ci vuole, care senatrici e cari senatori, un'operazione verità, a cominciare dalla verità per cui gli interessi cui gli interessi dell'Europa non potranno mai coincidere con quelli degli Stati Uniti e che chi sta pagando i costi sociali ed economici di questa guerra in termini di inflazione, di caro bollette e di crisi energetica sono i cittadini europei e i cittadini italiani, non quelli statunitensi. non quelli statunitensi. Questa guerra sta facendo male alle sue famiglie, presidente Meloni, e alle sue imprese. Non cerchi qui di diventare la protettrice perché sono le nostre imprese che stanno soffrendo in questo momento, non quelle che hanno piani di sostegno economico che lei ancora non ci ha portato. Lei deve venire qui non a farci bei discorsi, con la retorica dell'interesse nazionale e della libertà: lei deve dirci come intende darci da mangiare, come intende sfamare le fasce più deboli. *(Applausi)*. Certo, come ce ne ha dato mostra nella legge di bilancio, lei è bravissima a utilizzare i più vulnerabili e i più fragili come bancomat; lei è bravissima a tagliare il sostegno a tagliare il sostegno a chi è in difficoltà; lei è bravissima a non aggredire i privilegi di chi ha tanto, a discapito e detrimento di chi ha poco. Serve un'operazione sincerità, Presidente. Lei doveva venire qui per riferirci sinceramente lo stato dell'economia nazionale alla luce di questa crisi e portarci delle risposte, non farci discorsoni sull'interesse nazionale e sulla libertà. E allora, sincerità per sincerità, perché non ce lo dice? Lo abbiamo capito tutti, per cui squarciamo questo velo di ipocrisia: questa non è più la guerra tra Kiev e Mosca, questa è la guerra tra la Russia e la NATO e, se non la smettiamo di continuare a operare come una succursale della NATO, andremo incontro alla terza guerra mondiale. Ha letto le agenzie di questa mattina? Ha saputo delle esercitazioni aeree russe nell'*enclave* di Kaliningrad, tra la Lituania e la Polonia?

è una frase che disse Kennedy nel '62, con la crisi dei missili, sventando per un soffio la terza guerra mondiale. Non bisogna avere paura

che conviene ad altri, ma non ai cittadini europei, né men che meno ai suoi concittadini italiani.

Presidente Meloni, lei nei prossimi giorni andrà in Europa con un bel peso sulle spalle, il peso degli italiani e delle aspettative che gli italiani ripongono in lei. Mi sembra un peso importante, visto e considerato che fino a adesso in Europa non è andata a dire signorsì, ma a portare

ci venivano chieste determinate cose. Forse, Presidente, i colleghi del MoVimento 5 Stelle questa cosa non se la ricordano - ahimè - e bisogna ricordargliela tutte le volte. È giusto, Presidente, continuare a rafforzare il mercato unico europeo e adattarlo alle sfide che provengono da *competitor* internazionali sempre più forti, che aggrediscono con maggiori risorse l'attuale crisi, come gli Stati Uniti, o che spesso non rispettano le tutele dei lavoratori e i vincoli ambientali che abbiamo noi, come la Cina. Ma cosa vuol dire, Presidente e colleghi, tutelare il mercato unico europeo? Per noi della Lega significa anche tutelare i nostri prodotti tipici, il *made in* di qualità che contraddistingue l'Italia e altri Paesi europei nel mondo. E allora, colleghi, in un vero mercato unico non possiamo pensare di farci la guerra al nostro interno, con le etichette allarmistiche dell'Irlanda, con la carne e il latte sintetico, del Prosek, che non è ancora stato risolto, o quello dell'aceto balsamico, che siamo ancora qui ad aspettarle, o con iniziative strambe come quella del nutri-score, che si pongono l'obiettivo giusto e condivisibile di tutelare la salute dei consumatori, ma che tuttavia forniscono informazioni distorte che poco hanno a che vedere con la salute e molto con una battaglia commerciale scorretta e penalizzante per il nostro Paese. Su questo l'Italia dev'essere intransigente ai tavoli europei, trovando le giuste alleanze e sostenendo così una battaglia che potrà solo rafforzare la presenza commerciale europea nel mondo, grazie a una qualità di prodotti che il mondo ci invidia. Presidente, non le parlo della questione dei balneari, sarebbe troppo facile. È una questione che lei conosce, perché il vero nemico dei balneari non sta in Europa, ma in Italia, quindi sarà inutile andare a parlarne prima di aver risolto la questione in Italia, con i vari poteri dello Stato che prendono decisioni sempre più anomale. *(Applausi)*. L'Europa sta cambiando strada e noi non possiamo che esserne contenti. Sembra finalmente finita l'epoca dell'*austerity* e si affaccia la volontà di aprire una fase nuova, basata sulla crescita come strumento di benessere e maggiore stabilità finanziaria. Va bene quindi la discussione che si sta facendo sul nuovo Patto di stabilità, sulla scia di quanto già abbiamo visto con il *recovery plan* all'indomani della pandemia. Le nuove condizioni che si sono create con l'aumento dei costi delle materie prime e la crisi energetica seguita all'invasione russa dell'Ucraina ci spingono però a essere più pragmatici e, al tempo stesso, più ambiziosi. Certo, dovremo dare agli Stati europei più possibilità di investire nella crescita e nella transizione energetica e digitale, consentendo una maggiore flessibilità nei piani di rientro del debito pubblico, ma non possiamo guardare al futuro ignorando quello che abbiamo a disposizione nel presente. presente. Questa discussione deve coinvolgere anche gli strumenti che l'Europa ha già messo in campo, tutti gli strumenti. Fa bene allora la presidente Meloni a chiedere una riflessione vera e approfondita sulla funzione del Oggi l'Italia viene accusata di bloccare quel fondo, ma in realtà quello che chiediamo è di guardare avanti e di prendere atto che la sua funzione e i vincoli che esso impone sono ormai superati. Se quella del MES non è una battaglia di retroguardia, ma di prospettiva, la stessa cosa vale anche per gli obiettivi di efficientamento e transizione energetica. Non pensiamo che sia sbagliato migliorare l'efficienza energetica delle nostre case o ridurre le emissioni provocate dalle automobili. Sono obiettivi che condividiamo e sosteniamo da sempre. Diciamo una cosa diversa: non possono essere cittadini e imprese a sostenere sulle loro spalle il peso di tutto questo percorso. Servono risorse europee, europee, realismo nei tempi di realizzazione e più attenzione alle specificità dei singoli Paesi. L'Europa è un insieme di singoli Paesi, non siamo tutti la stessa cosa. Più atti concreti e meno demagogia: purtroppo, da parte di chi ci gestisce in Europa - e non penso solamente alla parte politica, ma soprattutto ai tecnici che ci sono in Europa - vedo tanta demagogia e poco pragmatismo. Noi oggi rischiamo di passare da una dipendenza all'altra: abbiamo conosciuto la dipendenza dal petrolio, che ci ha costretti a un duro periodo di *austerity* negli anni Settanta; stiamo provando a uscire dalla dipendenza dal gas russo e va dato atto a questo Governo - e anche a quello precedente - di aver lavorato bene per superare una fase difficilissima e tornare così, pian piano, a ridurre i costi dell'energia. Stiamo attenti, perché non è finita qui: dobbiamo insistere nel differenziare il più possibile le fonti energetiche e nel potenziare la produzione italiana di energia da fonti rinnovabili, per evitare che l'instabilità di altri Paesi produttori ci travolga nuovamente. Oggi dobbiamo fare in modo che le nostre scelte non ci portino dritti verso un'altra dipendenza, quella da materiali come il litio e dalla produzione di batterie, che si concentra soprattutto in Cina. *(Applausi)*. Diciamolo chiaramente: tutto questo ci renderà dipendenti dalla Cina. Per questo chiediamo all'Europa più prudenza nell'abbandonare la produzione di motori a combustione. Il commissario Timmermans nei giorni scorsi ha garantito il rispetto del principio della neutralità tecnologica; quello che gli chiediamo è di passare dalle parole ai fatti. Ancora una volta, vogliamo cose concrete. Consentiamo e sosteniamo la ricerca e la produzione di carburanti alternativi: così possiamo insieme ridurre le emissioni, fino ad azzerarle, ed evitare di finire schiavi del regime di Pechino. Infine, Presidente, la tragedia di Cutro non può essere dimenticata dall'Europa, né può essere ridotta a un problema esclusivamente italiano. Ha fatto bene la presidente Meloni a scrivere immediatamente alla presidente von der Leyen e a chiedere un preciso impegno della Commissione europea in tema di migranti. Troppe volte - l'abbiamo sentito nella XVII, così come nella XVIII legislatura - siamo stati lasciati soli (e ancora oggi lo siamo) a difendere le nostre coste, che - ricordiamolo - sono i confini europei, a salvare le persone abbandonate in mare e a combattere i trafficanti di esseri umani. L'Europa deve prendere atto che quanto ha fatto finora non basta; non bastano più le parole, non bastano più gli incontri, non basta più vedere *leader* europei che si abbracciano e promettono e basta. Dopo il drammatico terremoto in Turchia, quell'argine a Est non regge più. La barca affondata nello Ionio ha attraversato mezzo Mediterraneo e quelle persone avevano visto a lungo le coste europee prima di arrivare in Italia. Non basta più la segnalazione di un elicottero, serve un impegno diretto dell'Europa nel Mediterraneo. Cosa ci faceva quella barca in mezzo al Mediterraneo, senza che nessuno abbia detto niente? *(Applausi)*. Chiediamolo ai colleghi della Grecia, a Cipro e all'Europa: perché quella barca ha attraversato mezzo Mediterraneo per arrivare in Italia e poi l'Europa ha incolpato noi? Serve un nuovo patto europeo che definisca come comportarsi con i richiedenti asilo e con i migranti economici, redistribuendo i primi e facilitando gli accordi di ingresso per i secondi, sulla base di quote definite a livello nazionale. Per gli altri mi dispiace, ma non ci può essere posto, perché, al contrario di quanto vorrebbe far credere qualcuno, non basta accogliere, ma serve anche integrare. E, se non c'è lavoro, non può esserci integrazione; se non c'è lavoro per gli italiani, non può essercene per gli altri. Se non c'è integrazione, crescono il disagio sociale, l'insicurezza e l'illegalità. In questo l'Europa può e deve fare molto di più, sostenendo gli accordi bilaterali per prevenire le partenze irregolari, combattere gli scafisti, facilitare i rimpatri e creare corridoi d'immigrazione legale. Oggi, signor Presidente, signora *Premier*, il Papa ha parlato di diritto a non dover emigrare. lo ha detto il Papa, non il *leader* della Lega: il diritto a non dover emigrare. Quel diritto devono averlo tutti coloro che scappano da guerre o persecuzioni. Gli afgani, quelli che sono morti a Cutro, che scappano dal quel Paese, scappano da una situazione che abbiamo creato noi occidentali, colleghi, non dimentichiamocelo. Siamo noi che siamo scappati dall'Afghanistan, li abbiamo abbandonati. nelle mani dei talebani. Le donne e i bambine afgani devono essere aiutati, come abbiamo fatto per le donne e per i bambini ucraini. Presidente Meloni, noi ci fidiamo di lei. Gli italiani si aspettano di essere degnamente rappresentati in Europa.

un'agenda molto fitta, ricca di temi molto importanti per il futuro dell'Europa e del nostro Paese. Io mi concentrerò su due nodi due nodi a cui la presidente Meloni - che spero non me ne vorrà - credo abbia dedicato meno tempo di quanto meriterebbero: l'energia e la transizione ecologica sono il primo e la riforma della *governance* economica dell'Unione è il secondo. Sul primo punto credo che tutti debbano riconoscere che i mesi passati hanno visto passi in avanti molto significativi in materia di energia, di scelte per accelerare la transizione ecologica: da dicembre c'è il *price cap* sul petrolio russo; da febbraio c'è il meccanismo di correzione del mercato del gas; la Commissione ha presentato pochi giorni fa la proposta di riforma dell'assetto del mercato elettrico, la Banca europea dell'idrogeno, il *Net-zero industry Act* e il *Raw material Act*, per ridurre la dipendenza da materie prime essenziali; è poi in discussione l'importantissimo regolamento sul *phaseout* al 2035 della produzione di automobili con motore endotermico. Ora, abbiamo ascoltato con attenzione l'intervento della presidente Meloni e l'avvio di questo dibattito. Differenziandoci in questo dalle valutazioni che abbiamo ascoltato dalla Presidente e da altri colleghi, noi crediamo che mai come oggi perseguire la sostenibilità ambientale e la decarbonizzazione coincida largamente con la sostenibilità economica e sociale e con la sicurezza geopolitica del nostro Paese. Mai come oggi decarbonizzare vuol dire tagliare le bollette per le famiglie e per le imprese, proteggere l'economia e i posti di lavoro del nostro Paese. Mai come oggi ridurre e azzerare la nostra dipendenza dai combustibili fossili vuol dire rafforzare la sicurezza, l'affrancamento del nostro Paese dai regimi dittatoriali da cui oggi ci riforniamo di combustibili fossili. Certo, servono passi in avanti importanti, sono oggetto della discussione del Consiglio. La riforma del mercato dell'energia elettrica è cruciale per accelerare la transizione verso le rinnovabili, ma anche cambiare i meccanismi di formazione del prezzo, superando le distorsioni che abbiamo subito nei mesi della crisi energetica. Serve ragionare su nuovi strumenti di finanziamento pubblico e privato, perché serviranno investimenti enormi per la transizione verde. È necessario rafforzare le competenze e quindi investire nella scuola, nell'università e nella ricerca. Servono politiche, a livello europeo, ma anche nazionale, di accompagnamento. Faccio l'esempio più importante: il comparto dell'*automotive*, molto rilevante per l'economia italiana, pesa parecchi punti di PIL, fornisce centinaia di migliaia di posti di lavoro e costituisce un segmento rilevantissimo per la vocazione manifatturiera del nostro Paese. Il Governo in Europa, in Europa, come ha ribadito anche la presidente Meloni, sta dicendo no alla scelta del *phaseout* nel 2035, sì alla neutralità tecnologica e allo sviluppo anche dei *biofuel*. Vede, Presidente, io credo che il concetto di neutralità tecnologica in astratto sia condivisibile. Il presidente Deng, a proposito di Cina, diceva che non è importante il colore del gatto, purché prenda il topo; il nostro obiettivo dev'essere la decarbonizzazione, quindi la neutralità tecnologica in sé, in astratto, è un concetto condivisibile. Il punto però è capire da che parte sta andando il mondo e qual è oggi nel concreto la tecnologia più matura per decarbonizzare il settore dei trasporti. Vedete, il motore elettrico può piacere o non piacere, ha sicuramente dei limiti, ma ha anche dei pregi: oggi è la tecnologia più matura per andare verso emissioni zero nel settore dei trasporti; non a caso, la Cina, gli Stati Uniti e i grandi produttori stanno andando in quella direzione e anche i produttori europei, che usciranno prima del 2035 dai motori a combustione interna, stanno direzionando verso l'elettrico i loro investimenti. Dobbiamo allora dare certezze ai produttori e ai consumatori e, se il mondo sta andando in una determinata direzione, credo sia una pericolosa illusione coltivare il sogno che si possa andare in una direzione diversa. diversa. Dobbiamo prepararci invece a reggere e a difendere la nostra vocazione manifatturiera nell'*automotive* e i nostri posti di lavoro, tenendo conto con realismo di dove sta andando il mondo. Quanto alla *governance* economica, negli anni della crisi del debito sovrano sono emersi con forza i limiti di quella a livello europeo: il carattere prociclico delle regole, la mancanza di flessibilità, l'ottica di breve termine e il carattere stesso degli indicatori utilizzati, non osservabili e poco trasparenti. trasparenti. Crediamo che la proposta presentata dalla Commissione a novembre, con i piani differenziati, l'ottica di medio-lungo termine, la spesa netta come variabile chiave, siano un passo in avanti vero per superare gran parte di quei limiti. Mi sarebbe piaciuto ascoltarlo anche dalla presidente Meloni, ma credo che l'Italia debba ringraziare il commissario Gentiloni per il lavoro fatto per cambiare le regole di austerità che hanno complicato la vita agli italiani e agli europei. Certamente servono passi in avanti ulteriori e noi li indichiamo nella nostra proposta di risoluzione: escludere dalla spesa netta le spese per le riforme e gli investimenti, della *golden rule* per la quale dobbiamo batterci, perché l'Europa ha bisogno di enormi investimenti per la transizione ecologica e digitale e le regole di bilancio non devono ostacolare, ma anzi devono favorire un gigantesco piano di investimenti a livello europeo e nazionale. Abbiamo bisogno di flessibilità dei piani nazionali e di tenere conto delle specificità nazionali, quando si discute di stabilizzatori automatici da escludere dalla spesa netta. Varrebbe la pena di fare un ragionamento separato sul debito Covid, perché nel periodo 2020-2021 il cataclisma economico che ha investito l'Europa e ha costretto i Governi a rispondere opportunamente, facendo *deficit* e debito, è un evento eccezionale, che meriterebbe un percorso di rientro specifico. Abbiamo bisogno in Europa di meccanismi europei di stabilizzazione automatica, sul modello di Sure, che è stato un programma di successo (credo, signor Presidente, che almeno su questo siamo tutti d'accordo). Abbiamo bisogno di favorire una capacità fiscale dell'eurozona, per intervenire in circostanze eccezionali, e di avviare - ma questo richiede una revisione dei trattati

delle dinamiche economiche e di finanza pubblica, nei Paesi avanzati. Signor Presidente, queste sono le nostre proposte, perché difendere l'interesse nazionale - uso le parole della presidente Meloni - è un obiettivo che ci unisce, in quest'Aula e nel Paese. Quella che non condividiamo è la strategia che state seguendo per difendere l'interesse nazionale, perché, signor Presidente, riteniamo che affrontare l'emergenza climatica sia difendere l'interesse nazionale e che evitare o ridurre i danni della siccità, dello scioglimento dei ghiacciai e degli eventi climatici estremi sia interesse nazionale. Voi in Europa state dicendo di no a qualunque cosa venga avanti per accelerare la transizione energetica ed ecologica. Peraltro, state affrontando questa discussione - me lo permetta, signor Presidente - con un quadro di alleanze che secondo noi rende l'Italia più debole nel negoziato in Europa. In compenso, non state facendo nulla... l'Italia alla transizione che arriverà, nulla per aiutare l'*automotive* a riconvertirsi, nulla per accelerare la rigenerazione degli edifici. Anzi, avete smontato quel poco o tanto che c'era, a partire dal superbonus. Non fate alcunché per aiutare i lavoratori a reggere gli effetti e le conseguenze della transizione accelerando la creazione di lavoro. Questa non è una strategia: è qualcosa è qualcosa che rischia di portarci su un binario morto. È per questo, Presidente, che chiediamo al Governo di cambiare rotta: non per un obiettivo astratto, ma per difendere al meglio gli interessi nazionali del nostro Paese.

Onorevole Presidente del Consiglio, abbiamo ascoltato in questi minuti la sua esposizione sul prossimo Consiglio europeo, sul prossimo Consiglio europeo, che sarà incentrato su tre delle più grandi sfide che non soltanto questo Governo, ma il nostro Paese messo insieme, nella sua interezza, e l'Europa stanno affrontando nella loro storia.

Su queste tre sfide, su questi tre problemi credo che siano molti i colleghi in quest'Aula e in generale nel Parlamento italiano che hanno avuto modo e hanno consuetudine di contatti quotidiani o quasi con interlocutori parlamentari, di Governi, di entità, di ambienti economici stranieri.

e incoraggiamento all'Italia e al Governo Meloni che è costante. È un elemento costante di tutti gli incontri e le interlocuzioni che abbiamo con esponenti di Paesi occidentali, europei o di altre realtà geopolitiche. Dicevo fiducia nell'Italia. Questa dovrebbe essere una costante nell'attività dell'intero Parlamento, Parlamento, anche dei partiti di opposizione, oltre che della coalizione che sostiene il Governo. Dovrebbe essere un obiettivo costante promuovere la fiducia nell'Italia e la credibilità del nostro Paese e degli italiani come principio fondamentale del nostro interesse nazionale; dovrebbe essere una missione - come si dice - per ogni eletto dal popolo italiano che siede in quest'Aula. E in effetti questo è avvenuto in tantissime stagioni della nostra storia repubblicana. È avvenuto negli ultimi trent'anni quasi costantemente, quando crisi di questa ampiezza si profilavano all'orizzonte; certo, con alcune significative eccezioni, ma è stato frequente l'appoggio anche di segmenti esterni alle maggioranze di Governo

da espressioni così polemiche e negative come quelle che abbiamo sentito? Credo che non ci sia niente che dimostri la realtà nella quale stiamo vivendo come il vertice che sta proseguendo in queste ore fra il presidente Xi Jinping della Repubblica popolare cinese, segretario del Partito comunista cinese, e il presidente Putin. In questo vertice è stato subito riaffermato come fra i due Presidenti ci sia un obiettivo condiviso: dettare le regole della nuova sicurezza europea e della sicurezza globale e riportare il mondo a una sorta di dominazione di volontà alternative, di poteri alternativi, che non sono quelli sui quali si basa il diritto internazionale. Sfortunatamente, queste espressioni e questi impegni vengono da due Presidenti che sono l'incarnazione stessa di regimi totalitari, negatori della nostra libertà, alternativi ai nostri valori. alla prima questione, l'Ucraina, c'è un'assoluta urgenza di ristabilire una narrativa ed è urgente combattere contro la disinformazione che viene alimentata non soltanto dai due Paesi che ho citato, ma anche all'interno dell'Europa dai nostri Paesi, da voci che automaticamente si schierano su delle narrative negatrici di fatti e delle realtà più evidenti. Ricordiamo i figuranti di Bucha. Ricordiamo i motivi dell'entrata in guerra della Russia che sostiene di esser stata aggredita, perché è stato aggredito il Donbass, territorio ucraino riconosciuto da tutti. ricordiamo tante altre cose nelle quali c'è una congiunzione astrale fra le teorie propalate da due Presidenti che ho citato, ma purtroppo anche da diverse forze politiche del nostro Paese e da diversi amici di quei due sistemi. quindi contrastare la propaganda, riportare una narrativa. Si sta facendo molto in Europa. Ma, se c'è una cosa su cui il Governo italiano è impegnato e credo che stia acquisendo anche la comprensione di altri Governi europei e delle istituzioni comunitarie, è su questi punti.

Ci si deve guardare anche da delle presentazioni ipercritiche, come quelle di cui sono stato testimone in una recente riunione a Bruxelles con istituzioni parlamentari e servizi della Commissione al Parlamento europeo,

per contestare il quale potevamo parlare soltanto per novanta secondi. Queste sono le norme del confronto e le costruzioni alle quali siamo sottoposti quando si parla d'Italia e delle rappresentazioni sull'economia italiana. La terza sfida di proporzioni gigantesche riguarda le migrazioni. Non c'è dubbio che gli ultimi passaggi

contenuti in un documento importante, che è la lettera di ieri del presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che costituisce la sintesi delle cose che lei ci ha spiegato e che verranno discusse dopodomani.

strategie di sviluppo di fondamentale rilevanza, il piano Marshall per l'Africa, evidentemente unite a strategie anche di radicamento della legalità di Stato di diritto e di diritti umani in quei Paesi. È la mancanza di questi elementi fondamentali a creare le distorsioni di base nella possibilità di creare occupazione e anche volontà di rimanere da parte delle persone che altrimenti emigrano e creano una massa in uscita verso l'Europa. Dobbiamo guardare anche alle problematiche della sicurezza. Ricordiamoci ad esempio che il Concetto strategico della NATO del 2022 indicava già con precisione, grazie proprio agli interventi della Spagna e dell'Italia, la necessità di contrastare decisamente le crescenti interferenze straniere negli Stati africani. E di questo lei, onorevole Presidente del Consiglio, ha parlato in questa occasione. L'Italia, l'Europa e l'Occidente hanno il coraggio, la determinazione

Signor Presidente, sarò abbastanza breve e ovviamente intendo replicare soprattutto alle cose che non condivido. Quindi non me ne vorranno i senatori di maggioranza - tendenzialmente ho condiviso i loro interventi - se mi concentrerò di più su quello che ho sentito dire dall'opposizione. Mi pare che, anche seguendo che, anche seguendo la relazione che avevo fornito all'Assemblea, siano sostanzialmente tre le questioni sulle quali si sono concentrati gli interventi durante il dibattito: il tema delle migrazioni, il tema della transizione ecologica e il tema del conflitto Mi corre l'obbligo di dare alcune risposte in base a quello che ho sentito dire. Confesso che sul tema dell'immigrazione continua a non essermi chiaro quale sia la proposta che arriva dai banchi Ho sentito, ad esempio, il collega Lorefice dire che occorre sicuramente fermare gli scafisti, cooperare con l'Africa e lavorare sui decreti flussi. Temo che sia esattamente quello su cui il Governo lavora. Abbiamo infatti presentato una serie di norme che vogliono colpire il traffico di esseri umani. Contemporaneamente abbiamo avviato, soprattutto a livello europeo, un dialogo e una proposta che da una parte lavora lavora sull'aspetto securitario, ma che ha nel suo elemento fondamentale un diverso rapporto tra l'Europa e i Paesi africani. Abbiamo noi stessi lanciato quello che voi ormai conoscete come piano Mattei per l'Africa, andando in giro in lungo e in largo per tutta l'Africa a cercare di portare investimenti, chiedendo anche all'Unione europea di darci una mano a investire.

grazie a un approccio non predatorio, come quello che oggi vediamo in molti Paesi africani a causa soprattutto dell'assenza dell'Europa, ma da pari a pari che vuole portare investimenti, lavoro e formazione.

È l'Italia che negli ultimi anni ha azzerato i decreti flussi, perché tutte le quote di immigrazione possibili erano coperte da chi entrava illegalmente. *(Applausi)*. Questa Nazione in sostanza diceva che chi voleva entrare in Italia lo poteva fare solo mettendosi nelle mani degli scafisti. È questa secondo me è una cosa totalmente irragionevole. Noi, quindi, mentre facciamo del nostro meglio per fermare gli scafisti, riapriamo i decreti flussi, li immaginiamo triennali, cioè diamo una certezza e una prospettiva a chi vuole venire in Italia legalmente, e lavoriamo con i Paesi del Nord Africa per portare investimenti e sviluppo, sperando anche che si possa mettere insieme la formazione che si può fare da noi e il lavoro che eventualmente si può fare qui o tornare a fare nei propri Paesi d'origine. Mi pare un ragionamento sensato, a fronte del quale non rilevo grandi proposte

giorno. Segnalo sommessamente che siamo oggettivamente di fronte a un fenomeno che oggi assume una portata che non aveva in passato, per temi che sono variegati, che voi conoscete meglio di me e che non elenco per ragioni di tempo. di tempo. Oggi abbiamo un problema enorme legato alla stabilità e a un possibile *default* della Tunisia che non si riesce ad affrontare perché il Fondo monetario internazionale, che aveva avviato una trattativa con la Tunisia per sostenerla, a un certo punto l'ha bloccata. la stessa Commissione europea - ho parlato ieri con il commissario Gentiloni, che aveva immaginato già all'inizio di questo mese di recarsi in Tunisia per cercare di affrontare la vicenda - ha poi rimandato il viaggio bilaterale e l'iniziativa. quindi, fa del suo meglio parlando con tutti gli omologhi possibili e immaginabili per cercare di sbloccare uno stallo che - a mio avviso - non ci aiuta e che rischia di peggiorare drammaticamente la situazione. Grazie per averlo ricordato, quindi, ma è esattamente il lavoro che noi facciamo

Le dirò che la mia coscienza è perfettamente a posto *(Applausi)*. Spero che sia a posto anche la coscienza di chi usa le morti di povera gente per fare propaganda.

profonda la sua accusa dice, citando Pasolini, che tutti sappiamo ma non abbiamo le prove. Questa è l'idea di giustizia che in questa Nazione hanno alcuni, perché nello Stato di diritto sono le prove che fanno un colpevole, non sono i colpevoli che definiscono le prove.

quando l'Italia viene lasciata da sola ad affrontare un problema che da sola non può affrontare, sfuggirà sempre qualcosa, ci sarà sempre qualcosa che andrà storto - vi rendete conto di come vanifichiamo, anche ai fini delle risposte che ci servono,

Ancora la collega parlava di Visegrad, che vuole alzare i muri, che non vuole partecipare alla redistribuzione dei profughi. Credo che vada un po' aggiornato il manuale degli *slogan*, perché i Paesi di Visegrad oggi (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia) stanno accogliendo milioni di profughi ucraini *(Applausi)* e lo stanno facendo da soli. E, se alcuni che sento qui partecipassero alle riunioni del Consiglio europeo, scoprirebbero che, per esempio, tra quelli che chiedono muri per fermare l'immigrazione illegale c'è il Governo austriaco, la cui maggioranza è formata da esponenti del Partito popolare europeo e dei Verdi. Temo, quindi, che la situazione non sia semplice come invece la fanno alcuni e che si debba capire che è un problema che impatta su tutta l'Europa, che ogni Nazione cerca di risolvere nel migliore dei modi, ma sul quale ovviamente noi dobbiamo lavorare per raggiungere le soluzioni migliori possibili anche per i confini marittimi - come dicevamo - che sono molto particolari e che rendono la questione più complessa. Quanto

Il senatore Licheri, poco dopo, ha denunciato il rischio di una tassa patrimoniale figlia delle scelte della Banca centrale europea. Le due cose si possono mettere insieme, perché temo che si debba spiegare, colleghi del MoVimento 5 Stelle, che la direttiva sull'efficientamento energetico degli edifici rischia di diventare una tassa patrimoniale sugli italiani. *(Applausi)*. Quando in Europa abbiamo chiesto: «Scusate, ma come si sostiene? Ci sono dei fondi dedicati all'efficientamento?», Peccato che i primi provvedimenti per l'efficientamento energetico delle case vadano conclusi entro il 2027. È, quindi, in questo caso forse si deve spiegare agli italiani che non potranno efficientare le loro case gratuitamente, ma dovranno pagare in una condizione già difficile e forse non ci conviene in questa fase aggiungere ulteriori problemi. È la ragione per la quale insisto nel dire che determinati obiettivi, che sono sicuramente condivisi dal Governo italiano, devono essere perseguiti con una sostenibilità di fondo, sia sul piano sociale, sia sul piano economico. Il senatore Misiani ha sostenuto che dobbiamo capire la direzione verso la quale sta andando il mondo. senatore, penso che sia finita l'epoca in cui l'Italia subisce i processi. Vorrei che questa Nazione, consapevole del suo ruolo, contribuisse a definire dove deve andare il mondo È esattamente quello che tentiamo di fare, perché poi in alcuni casi, quando con garbo abbiamo posto questioni che non erano solo problemi italiani, altri hanno hanno compreso le nostre posizioni e ci hanno dato una mano e probabilmente non lo avrebbero fatto, se l'Italia non avesse avuto il coraggio di porre la questione. Ciò non toglie che le alleanze si possono costruire su ogni materia. Anche qui il riferimento continuo ai nostri alleati giusti, ai nostri alleati sbagliati, temo che si debba tener conto del fatto che noi dialoghiamo con tutti, con tutti, perché difendiamo il nostro interesse nazionale: non viviamo mai la politica estera come un fatto di tifoseria, amico-nemico. Noi dialoghiamo con tutti, ragionando su come costruire sintesi in rapporto al rispetto per gli altri che difendono i loro interessi nazionali e alla difesa del nostro interesse nazionale. Si può fare tranquillamente e lo abbiamo visto, perché alcuni risultati che sono scritti sulle conclusioni dei precedenti Consigli europei sono figlie di questo lavoro. Ribadisco, quindi, che condividiamo gli obiettivi della transizione verde; condividiamo l'obiettivo di azzerare le emissioni di CO2 entro il 2035, ma rivendichiamo la neutralità tecnologica. È un tema legato al ruolo dell'Europa. L'Europa può stabilire gli obiettivi e stabilisce gli obiettivi, ma non è l'Europa che deve dirmi come raggiungo quegli obiettivi *(Applausi)*, perché io non cambio idea sul tema

che, sull'altare della decarbonizzazione, ci consegna diritti alla deindustrializzazione. Io penso che le cose vadano messe insieme. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo garantito il nostro sostegno agli obiettivi. Abbiamo rivendicato la neutralità tecnologica e non ci siamo limitati a spiegare le buone ragioni che ci portano a ritenere che la proposta di regolamento sulle emissioni di CO2 per i veicoli leggeri è inopportuna nella sua forma attuale, banalmente perché rischia di consegnarci a nuove dipendenze, come ho già detto e come tutti quanti sappiamo. Noi abbiamo illustrato, dati alla mano - e in questo evidentemente siamo stati convincenti - che è possibile conseguire lo stesso risultato, cioè gli obiettivi della transizione verde, impiegando tecnologie diverse rispetto all'elettrico, sulle quali oltretutto segnalo sommessamente che l'Italia rappresenta rappresenta anche un'avanguardia. Penso ai biocarburanti, ai carburanti sintetici, all'idrogeno. Noi vantiamo tecnologie di avanguardia su queste materie. Perché, piuttosto che lavorare per sviluppare le nostre tecnologie di avanguardia, vogliamo passare dalla dipendenza dal gas russo alla dipendenza dall'elettrico cinese? Io non riesco a capire. *(Applausi)*. Stiamo cercando di difendere l'interesse nazionale, lavorando su quello che ci può rafforzare economicamente e mantenendo gli stessi obiettivi, perché - ribadisco - sono materie pragmatiche e con pragmatismo le vogliamo le vogliamo affrontare.

abbiamo affrontato e stiamo affrontando la questione idrica, che è una grande questione. Abbiamo ereditato oggettivamente una situazione abbastanza complessa. Stiamo lavorando per istituire a Palazzo Chigi una cabina di regia con tutti i Ministeri interessati, perché vogliamo arrivare alla definizione di un piano idrico straordinario nazionale, d'intesa con le Regioni e con gli enti territoriali, perché si possano individuare le priorità di intervento e la loro adeguata programmazione, anche utilizzando nuove tecnologie e avviando una campagna di sensibilizzazione sull'uso responsabile della risorsa idrica. Il Governo sta lavorando a un provvedimento normativo urgente, che contenga le necessarie semplificazioni e deroghe per accelerare i lavori essenziali, e intende anche lavorare all'individuazione di un commissario straordinario che abbia poteri esecutivi rispetto a quanto definito dalla cabina di regia. Questa è una grande materia, che non rientrava ovviamente nei temi di oggi, ma, poiché è stata citata dai colleghi, ne ho approfittato per raccontarvi quello che il Governo sta facendo. Dopodiché, mi avvio alla conclusione.

relative al Consiglio europeo e, quindi, sono tenuta a parlare di quello che si discuterà nel Consiglio europeo. Poi, quando volete, vengo a parlare della situazione economica italiana. Si è parlato della guerra russa contro la NATO e della NATO contro la Russia.

Stelle, che prediligerebbero un'alleanza più stretta magari con la Cina rispetto ai Paesi NATO; partiti che auspicano una resa dell'Ucraina, sperando che questo possa allontanare il conflitto invece di avvicinarlo, come purtroppo sarebbe. Ma non è la posizione di questo Governo. *(Applausi)*. Su questo non ci capiamo. Noi non siamo di questo avviso. 5 Stelle per aggiornarli, come del resto già l'Italia ha potuto fare durante i Governi Conte, che hanno aumentato le spese militari sia in valori assoluti, sia in rapporto al prodotto interno lordo. Quindi, evidentemente, anche loro si rendevano conto di quanto questo fosse importante. forse è proprio questo il punto. C'è una politica che ha due facce: una in privato, nei consessi internazionali, quando bisogna cercare di trovare soluzioni, e una in pubblico, quando bisogna fare propaganda fare propaganda con i cittadini. La propaganda, per carità, la fanno tutti, però ci sono quelli che mettono la faccia sulle scelte che fanno. Io voglio rappresentare esattamente un Governo che mette la faccia su quello che fa. *(Applausi)*. Concludo dicendo quanto ho sentito dire che io andrei in Europa a prendere ordini. Guardi, questo lo vedranno i fatti, ma una cosa gliela dico: non mi vedrà mai vedrà mai - preferisco piuttosto dimettermi - presentarmi al cospetto di un mio omologo europeo con i toni con i quali Giuseppe Conte andò al cospetto di Angela Merkel *(Applausi)* a dirle che il MoVimento 5 Stelle erano ragazzi che avevano paura di scendere nei consensi, ma alla fine avrebbero fatto quello che loro chiedevano. Preferisco dimettermi che rappresentare una Nazione del genere.

del ministro Fitto e, quindi, del Governo, chiederei, ai sensi dell'articolo 102 del Regolamento, di poter votare per parti separate e preannuncio che per quanto riguarda

maggioranza. Sul resto, per quanto riguarda gli impegni sull'Ucraina, come è giusto che sia in un momento particolare e difficile dell'Italia e dell'Europa, noi saremo a sostegno della politica del Governo. PRESIDENTE. Senatrice Paita lei ha chiesto di votare per parti separate la però poi mi ha detto che voterà alcune parti della proposta di risoluzione di maggioranza. Quindi chiede di votare anche la risoluzione di maggioranza?

i temi oggetto della nostra discussione oggi in Parlamento sono l'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, la crisi energetica, la competitività delle nostre imprese nell'ambito del del Mercato unico europeo, la questione migranti. Tutto questo tocca la vita concreta di ciascuno di noi in quanto cittadini italiani ed europei. Sono temi sui quali sosteniamo convintamente la posizione del Governo. Parto dalla questione migranti; la politica per il controllo dei flussi migratori non può prescindere da un'azione dell'Unione europea nel quadro della politica europea di vicinato, prestando particolare attenzione ai Paesi del Nord Africa e supportando il processo di stabilizzazione dell'area del del Mediterraneo. I flussi migratori non sono e non possono essere un problema solo dell'Italia. La tragedia di Cutro ci insegna proprio questo; l'Europa non può e non deve voltarsi dall'altra parte. Come ha evidenziato lei, presidente Meloni, le frontiere marittime dell'Italia sono le frontiere di tutta l'Europa. Credo che sia servito proprio a questo lo scambio di lettere tra lei e la presidente della Commissione europea. Ricordo a tal proposito i progressi compiuti nelle conclusioni del vertice del 9 febbraio scorso, in cui si riconosce che la situazione migratoria è una sfida europea che richiede una risposta europea. In questo contesto riteniamo essenziale promuovere la cooperazione con i Paesi di origine e di transito per contrastare il *business* dei trafficanti di esseri umani, come consideriamo altrettanto fondamentale regolamentare i flussi di immigrazione legale verso l'Europa e superare in maniera definitiva quelli che sono stati i principi di Dublino, per arrivare ad un nuovo sistema basato su un adeguato bilanciamento tra i principi di solidarietà e di responsabilità. Così come consideriamo assolutamente cruciale difendere il lavoro di Guardia costiera, Guardia di finanza, Marina militare e le altre Forze dell'ordine che hanno sempre fatto il loro dovere; accusarli di non salvare è non solo ingiusto, ma anche un'operazione di propaganda inaccettabile e strumentale. Nell'ambito del Consiglio europeo si discuterà anche della situazione internazionale alla luce del conflitto in Ucraina. La sua recente visita a Kiev, Presidente, ha suggellato la posizione dell'Italia a fianco del popolo ucraino. Sulla politica estera, cari colleghi, si parla con una sola voce e non si possono lasciare spazi Su questo punto la maggioranza è da sempre rimasta compatta e coerente con le sue posizioni, al contrario di quanto purtroppo stiamo vedendo nelle opposizioni. A tal proposito vorrei ricordare la risoluzione delle Nazioni unite dello scorso febbraio, in cui l'Italia ha ribadito la propria posizione atlantista. Siamo dalla parte del popolo di Kiev e lavoriamo per una pace completa, giusta e duratura.

alla prospettiva della pace giusta. Ecco perché sosteniamo l'Unione europea, che continuerà a lavorare ad un piano di pace. Siamo altrettanto convinti che si debba sostenere, insieme a tutti gli altri Paesi membri, il processo di ricostruzione dell'Ucraina. presidente Meloni più volte ha parlato di un piano Marshall per l'Ucraina. Ecco perché sosteniamo il lavoro del Governo, che organizzerà il prossimo 26 aprile una Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, con il contributo delle imprese italiane. L'Europa che oggi è chiamata a svolgere un ruolo di primo piano in questo è anche l'Europa che nel secondo Dopoguerra, all'indomani di un conflitto mondiale, poneva le basi per un'unione politica ed economica che ha assunto le forme che oggi tutti noi conosciamo. Da oltre trenta anni, dal 1993, il mercato unico europeo è una realtà tangibile, su cui va disegnata una strategia di lungo termine. In materia economica ribadiamo la massima attenzione in favore della competitività delle nostre imprese, attraverso il pieno utilizzo degli strumenti dell'Unione europea appropriati e il ricorso all'uso flessibile dei fondi europei. Sui temi come Net zero industry act e la strategia per la competitività a lungo termine dell'Unione europea la nostra linea è chiara e nitida: ci vuole una soluzione che tenga conto di tutte le esigenze, certamente quelle del sistema produttivo e quindi dei lavoratori europei, ma anche quelle dell'ambiente. Industria e ambiente sono fattori che vanno a braccetto e non vanno contrapposti, l'uno dall'altro, come ricordava prima lei, signor Presidente. Ecco perché riteniamo, come maggioranza di centrodestra, importante e significativa la necessità di riconsiderare le politiche comuni a tutela della concorrenza, nel rispetto delle specificità industriali e sociali. La transizione verde e digitale del nostro tessuto economico, secondo noi, va rimodulata mediante un percorso che sia realmente sostenibile sul piano economico e sociale. Per fare questo occorre far sì che una rigenerazione in chiave *green* del patrimonio edilizio e la transizione *green* dell'*automotive* prendano in adeguata considerazione le esigenze e le specificità di Paesi come l'Italia. Pertanto riteniamo doveroso e sottolineiamo la linea del Governo sulla revisione completa della direttiva sull'efficientamento energetico degli edifici e sul settore dell'*automotive*. Si Si pone all'attenzione del prossimo Consiglio europeo anche il tema della riforma della *governance* economica. Serve un cambio di paradigma rispetto alle politiche di bilancio. Ciò che serve è un approccio realistico, flessibile, che consenta di individuare un percorso sostenibile di riduzione del debito e di controllo della spesa, senza però sacrificare l'importanza della crescita, delle politiche di coesione e degli investimenti. Ho apprezzato molto, signor presidente Meloni, un passaggio del suo intervento sulla crescita stabile e duratura, che è l'unica garanzia di riduzione del debito pubblico. Altro tema di estrema rilevanza è quello energetico. Siamo consapevoli che la sfida più importante per il sistema Paese è l'indipendenza e l'autonomia energetica dell'Italia. Ecco perché riteniamo assolutamente cruciale che a livello dell'Unione europea si lavori insieme con gli altri Stati membri ad una riforma dell'assetto del mercato dell'energia elettrica, affinché promuovendo sostenibilità e competitività si garantiscano prezzi dell'energia più bassi per imprese e famiglie e si favoriscano favoriscano gli investimenti sulle energie rinnovabili, in un'ottica *green* e di sostenibilità. Su questo tema, come sugli altri punti evidenziati nel suo intervento, il Governo e la maggioranza hanno un'idea chiara e precisa, che

ha affermato che questo non è il momento giusto per arrivare ad un compromesso tale da mettere fine alla guerra in Ucraina. Due giorni fa i *media* hanno parlato di indiscrezioni dal Pentagono secondo le quali gli Stati Uniti punterebbero su una grande offensiva a maggio con l'obiettivo di vincere la guerra. Ieri si è parlato di una nuova fornitura di armi da parte dell'Unione europea all'Ucraina quantificabile in due miliardi di euro, e da un anno sentiamo ripetere che non è il momento per ipotizzare una trattativa. Ecco, ci chiediamo quando quel momento arriverà, e se siamo realmente interessati a che arrivi. Ad oggi assistiamo all'opposto: a una *escalation* incontrollata, che ormai, Presidente, interessa direttamente anche il nostro Paese, perché mi meraviglio che non se ne sia nemmeno fatto cenno - la presenza in Italia di militari ucraini che qui si addestrano sfiora evidentemente lo stato di belligeranza. Dalla scellerata invasione russa fino a oggi i tentativi di seguire la strada della diplomazia da parte dell'Unione europea sono stati inesistenti e il suo Governo, presidente Meloni, mi pare si muova nella stessa scia silenziosa. Devo anche dire che trovo un po' singolare la totale mancanza di attenzione sua - ma innanzitutto dell'amministrazione americana - su quanto sta accadendo in questi giorni, cioè, sul cosiddetto piano cinese; non adesione, Presidente, ma almeno attenzione. Eppure, lo stesso presidente Zelensky aveva riservato un qualche elemento di interessamento. Un piano evidentemente insufficiente, anche ambiguo, su un tema importantissimo, naturalmente, decisivo dell'integrità territoriale dell'Ucraina, ma che meriterebbe - credo - un approfondimento diverso dall'essere invece cestinato senza appello che sia citato, non fosse altro per il fatto che è sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo, compresi quelli italiani. L'Italia e l'Europa sono giustamente a fianco dell'Ucraina fin dal primo giorno, ma hanno interpretato questo sostegno solamente come un atto militare, una reazione - mi verrebbe da dire - più che un'azione, a cui si accompagna, però, la totale sottovalutazione di quanto questo vero e proprio deserto diplomatico possa portare il mondo in un baratro devastante. È stato detto per mesi che l'invio delle armi fosse necessario per raggiungere un punto di equilibrio, che serviva un sacrificio grande per raggiungere tale obiettivo; è ora però di chiedersi quale sia l'obiettivo da perseguire con questi impegni e sacrifici. La domanda, Presidente, è questa: vogliamo la pace o vogliamo la sconfitta in campo aperto della Russia? Chiediamo che l'Ucraina sia libera, sicura e indipendente oppure che Putin sia arrestato e processato secondo il mandato di cattura internazionale emesso dalla Corte dell'Aia? Come vede, sono scenari non semplicemente diversi, ma profondamente alternativi. Personalmente credo che, dopo un anno di guerra, questa ambiguità vada risolta e chiarita. Credo che l'Unione europea avrebbe non solo il diritto, ma il dovere di chiedere chiarezza su questo punto e che l'Italia dovrebbe adoperarsi con ogni mezzo per spingere l'Unione in questa direzione, perché nell'alleanza atlantica il ruolo degli alleati non può essere solo quello di inviare armi e seguire le direttive. In questa crisi l'Europa è stata, purtroppo, inesistente. Non fatevi e non facciamoci illusioni: la guerra non sarà una parentesi, chiusa la quale tutto tornerà come prima. Se l'Europa non riuscirà ad avere una voce autonoma non esisterà come soggetto politico per lungo tempo. L'Unione europea deve prendere un'iniziativa politica; può chiedere con piena lealtà, ma anche con forza, che si convochi al più presto una conferenza multilaterale per la pace. L'Europa non solo può farlo, ma ha tutto l'interesse a spostare l'asse di questa crisi dalla ricerca della vittoria militare alla negoziazione multilaterale, come peraltro impone lo stesso Trattato dell'Unione. Ecco, credo che se non si tornerà a svolgere un ruolo politico gli anni futuri saranno molto difficili: vale per la guerra e per la pace, ma vale sempre, presidente Meloni. Questo Consiglio affronterà anche un altro tema di enorme importanza: la competitività dell'Europa sui mercati globali, un punto essenziale, tanto più nella fase difficile che stiamo attraversando. Purtroppo dietro questa formula si sono nascoste per anni le grandi ingiustizie del nostro tempo: la cancellazione brutale dei diritti dei lavoratori, la concentrazione della ricchezza in poche mani, l'impoverimento di massa. Nel nome della competitività si è imboccata la strada che ha portato l'1 per cento della popolazione a possedere i due terzi della ricchezza e che ha precipitato nella povertà 100 milioni di persone in Europa. Questa strada va abbandonata. Bisogna invertire la rotta, per esempio introducendo a livello di Unione europea un sistema di tassazione progressivo che permetta una effettiva redistribuzione della ricchezza, il contrario della *flat tax* che tanto vi piace, signora presidente del Consiglio Meloni, e che peraltro vi ha fatto definitivamente gettare la maschera. Altro che destra sociale; come vi ho detto tante volte, siete una destra liberista che sta penalizzando i più poveri e premiando i più avvantaggiati. redistribuire ricchezza, progressività fiscale ed anche una *governance* economica dell'Unione capace di imparare dagli errori del passato, archiviando per sempre quella formula fallimentare del rigore che invece alcuni ancora oggi, soprattutto nel Nord Europa, mirano a resuscitare. Nulla è più ingannevole e illusorio del miraggio di una competitività conquistata a spese e sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici; peraltro nessuno dovrebbe saperlo meglio di noi italiani, che per decenni abbiamo perseguito una strada basata sui bassi salari con gli effetti disastrosi che conosciamo. La diseguaglianza è diventata la cifra del nostro tempo; quella diseguaglianza che farete aumentare se non bloccherete lo scellerato progetto dell'autonomia differenziata, una scelta totalmente nefasta che penalizzerà profondamente un Meridione già in ginocchio

con l'illusione magari che per sgocciolamento - si dice così - si possano portare dei benefici anche al Sud. No, l'Italia ha bisogno di due motori per competere a livello globale, altrimenti a pagare il prezzo non sarà soltanto il Meridione, ma sarà anche lo stesso Nord, il cui destino sarà diventare il Sud povero e massacrato del Continente europeo. *(Applausi)*. Sta già accadendo; andatevi a guardare i dati del prodotto interno lordo e fermatevi prima che sia troppo tardi.

quanto ho già detto più volte in quest'Aula sulle immani responsabilità del suo Governo nei drammatici e recentissimi eventi, ma voglio fare un'altra considerazione. In queste settimane sono già emersi gli abituali conflitti tra egoismi nazionali, esattamente quello che non comprendete, esattamente la linea verso la quale sarete inevitabilmente destinati ad andare a scontrarvi: l'Italia che chiede all'Europa di farsi carico della difesa dei confini marittimi, i Paesi del Nord che chiedono all'Italia di impedire i cosiddetti movimenti secondari. È esattamente la stessa logica securitaria della fortezza assediata, alla quale si aggiunge ora anche quella del fermare le partenze, con l'aiuto però - lei non ne parla di Paesi come l'Egitto e la Libia. Chiedere aiuto ai Paesi che ignorano i diritti umani vuol dire legittimare gli assassini, vuol dire legittimare gli stupri, vuol dire legittimare i *lager*. Parlate di caccia ai trafficanti mentre finanziate la guardia costiera libica, quella che organizza il traffico degli esseri umani. Dite di voler allargare i flussi,

che dovrebbero essere per tutti quanti noi il primo obbligo politico ed etico. Dite che non possono farli le organizzazioni non governative, allora abbiate la forza di proporre in Europa

Italia, Germania e Francia come lati perfettamente in equilibrio di un triangolo alla guida dell'Europa. Cos'è rimasto nove mesi dopo? Che l'alleanza tra Parigi e Berlino guida e determina le scelte in autonomia. Non serve a niente lamentarsi se si viene esclusi, come nel caso del vertice a Parigi con Zelensky. L'autorevolezza bisogna guadagnarsela sul campo, ma è molto difficile farlo quando si promuove una visione retrograda del mondo, che avvicina Roma più ai Paesi di Visegrád che alle grandi capitali europee. Presidente Meloni, in campagna elettorale la parola da lei più pronunciata è stata "coraggio", ma sulla transizione ecologica, sulla gestione dei migranti, sui diritti civili questo Governo ha tutto fuorché una posizione coraggiosa. L'Italia è uno dei Paesi più colpiti dal cambiamento climatico: 13 miliardi di danni dalla sola siccità negli ultimi nove anni; una perdita annua del 10 per cento della produzione agricola; ingenti danni alle infrastrutture e alle abitazioni; 29 morti nel solo anno Mentre il presidente Mattarella lancia l'allarme e chiede un intervento corale a livello europeo, voi vi opponete a tutto quello che cerca di arginare la crisi climatica: vi opponete alla proposta europea per vietare la vendita di auto inquinanti dal 2035; vi opponete, insieme alla sola Polonia, alla direttiva per la riduzione dei consumi energetici delle abitazioni; siete l'unico Governo che nel Consiglio dei ministri dell'ambiente UE si oppone al testo per la riduzione delle emissioni industriali, tra le quali finalmente vengono incluse quelle da allevamenti intensivi. Per non parlare del vostro attivismo contro le alternative alimentari alla carne. Il vostro *leitmotiv* è che nulla deve essere toccato e tutto deve rimanere com'è. Purtroppo con questa filosofia non solo danneggiate il Paese, che ha tutte le potenzialità per abbracciare il nuovo modello di sviluppo, ma danneggiate anche la credibilità italiana. Questa opposizione al futuro non riguarda solo l'ambiente, ma purtroppo anche i diritti civili. Insieme ai vostri amici di Visegrád, avete detto no al regolamento di genitorialità transfrontaliera. Dimostrate una vera e propria ossessione per la maternità surrogata, che riguarda solo una piccola parte dei casi ed è pienamente lecita e regolamentata in tanti Paesi, anche europei. Le parole di uno dei vostri esponenti sulla maternità surrogata, definita come peggiore della pedofilia, si commentano da sole. Cercate di colpire gli omosessuali, ma a ricorrervi sono soprattutto le coppie eterosessuali. Inoltre, come ha più volte sentenziato la Corte europea, l'interesse del minore deve essere in ogni caso prevalente. Sui migranti, la vostra costante lamentela di non ottenere il sostegno dall'Unione è solo parte della storia, perché l'Italia è soprattutto un Paese di transito e l'Europa, a sua volta, si lamenta da sempre per l'assenza di controlli e per la facilità con cui i migranti vengono fatti uscire per raggiungere gli altri Paesi europei. Infatti le richieste di asilo

Meloni, ha menzionato l'Austria come esempio negativo, le vorrei dare una notizia: l'Austria, in relazione alla propria popolazione, è al secondo posto per quanto riguarda le richieste di asilo. Allora, se voi non rispettate i patti, è difficile che gli altri Paesi diano una mano nella redistribuzione. Inoltre, vicende come quella di Cutro o il decreto contro le ONG non aiutano di certo a migliorare il giudizio nei confronti dell'Italia perché, come sottolinea la ministra tedesca Baerbock, la priorità assoluta è salvare le vite nel Mediterraneo. E anche sul MES l'essere l'unico Paese che non lo ratifica, e quindi lo blocca a tutti, non è una buona idea, soprattutto quando si ha bisogno di tempo per il PNRR, del sostegno della BCE per l'acquisto dei titoli di Stato e di un nuovo patto di stabilità che superi i vincoli stringenti del passato. Presidente Meloni, non è vero che l'Italia ha tutte le carte in regola per esercitare un ruolo da protagonista. Il vostro approccio non è quello di un Paese fondatore dell'Unione, di una grande democrazia liberale, ma è specchio di un progressivo arretramento culturale che spinge l'Italia a perdere d'importanza e di valore. La domanda da farsi è soltanto una: quanto volete che l'Italia conti in futuro? Se volete un Paese all'altezza della sua storia, con una voce, come lei dice, sempre più ascoltata in Europa, cambiate sulla gestione dei diritti e sulle sfide imposte dal riscaldamento globale; se immaginate, invece, un Paese condannato a un costante e progressivo declino, allora non cambiate nulla: le state indovinando tutte, dalla prima all'ultima.

primo fra tutti, ovviamente, la guerra in Ucraina, un argomento sul quale non mi soffermerò nel mio intervento. Riteniamo infatti che vi sia una sola linea possibile: andare avanti a sostenere gli ucraini finché la Russia non accetterà di sedersi a un tavolo di trattative impegnandosi contestualmente per il ritiro totale e immediato dai territori aggrediti. Questa rimane l'unica strategia efficace per tenere in sicurezza l'Unione europea da nuove rivendicazioni del Cremlino e da ulteriori conflitti. Questa linea, adottata all'indomani dell'invasione russa da Mario Draghi e da lei portata avanti con coerenza, è la nostra linea. Continueremo dunque a sostenerla insieme ai provvedimenti conseguenti e speriamo che si comporteranno così le altre opposizioni responsabili. Allo stesso modo, voteremo a favore delle parti della risoluzione di maggioranza concernenti la tutela del mercato unico, l'energia e la necessità di rimodulare la transizione ambientale per evitare la desertificazione industriale dell'Unione europea. Voteremo invece contro il punto sulla *governance* economica per la vostra assurda ostinazione a non voler ratificare il MES e contro quello che mira a giustificare la vostra posizione sulle concessioni balneari. Quello che non abbiamo trovato nell'ordine del giorno del Consiglio, onorevole Presidente, è un punto formale specifico sulle migrazioni e anche nella risoluzione di maggioranza troviamo solo accenni generici a questo tema. Anche le bozze di conclusioni del Consiglio che stanno circolando sono vaghe e indefinite. Vorrei dunque cogliere l'occasione della sua presenza qui prima del Consiglio europeo per proporre alle forze politiche di maggioranza e opposizione una piattaforma concreta per affrontare il tema dei migranti. Mi è chiaro che la questione migranti è stata la più divisiva degli ultimi dieci anni, ma dovrebbe essere oggi altrettanto evidente che l'approccio ideologico fondato sulla contrapposizione porti aperti - porti chiusi non ha portato a nulla. Nel tempo sono caduti sia gli *slogan* relativi ai blocchi navali, sia quelli che promettevano accoglienza per tutti. La prova del Governo, a destra come a sinistra, ha smontato le soluzioni semplici, buone per i *talk show*, ma contemporaneamente ha lasciato intatto il problema. Siamo tutti - o dovremmo esserlo - in cerca di soluzioni praticabili, umane, razionali. L'abbandono delle rispettive inconcludenti posizioni a destra e a sinistra è reso necessario dal peggioramento del quadro umanitario. Già nel 2022 Frontex ha rilevato un aumento del 64 per cento degli arrivi e i dati del Ministero dell'interno rilevano come gli sbarchi siano triplicati. Lei ha chiesto un'opposizione corretta, seria e ponderata: non voglio neppure immaginare che cosa avreste potuto dire e fare, se oggi, invece di essere sui banchi del Governo, foste stati all'opposizione, signora Presidente. Colleghi senatori, possiamo decidere di passare i prossimi mesi ad accusarci gli uni con gli altri o prendere atto che non è il colore del Governo a determinare le emergenze migratorie e che non è sbandierando durezza o retoriche di segno opposto che si risolvono i problemi.

è parte integrante dell'identità italiana che volete preservare. Mettere le ONG in condizione di operare con meno efficacia è una decisione assurda, così come sostenere che quanto accaduto a Cutro è frutto di una pura casualità e che tutta ha funzionato come doveva. Gentile Presidente, se 88 persone muoiono a 40 metri dalle nostre coste, nulla ha funzionato come doveva. *(Applausi)*. Ammetterlo è doveroso, signora Presidente, tanto quanto evitare di insinuare che il Governo abbia deliberatamente fatto affogare uomini, donne e bambini. C'è una via di mezzo in cui si può dire qualcosa non ha funzionato e che si fa una bella indagine interna, cercando di capire come migliorare i processi? *(Applausi)*. Dobbiamo poi impegnarci per ripristinare totalmente una missione europea sul modello di Sophia per estendere l'area di pattugliamento, disporre di maggiori mezzi rispetto a quelli esclusivamente italiani di Mare nostrum. In cinque anni Sophia ha salvato 40.000 naufraghi, prima della scellerata decisione di Matteo Salvini di farla chiudere. quello per cui non esiste alcuna possibilità di accogliere indiscriminatamente chiunque voglia venire in Italia. Siamo il primo approdo per un Continente di 1,3 miliardi di persone, che crescerà 1,3 miliardi di persone, che crescerà nei prossimi quindici anni di altri 700 milioni e non possiamo contare sulla crescita economica, perché i migranti si muovono quando escono dalla condizione di povertà assoluta e hanno un minimo di disponibilità che li spinge a partire. Il terzo principio è conseguente al primo: le rotte di immigrazione illegale vanno chiuse e per farlo occorre implementare quello che presentammo all'epoca - io ero il rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, Renzi era presidente del Consiglio - il varo di un Migration compact che ha l'obiettivo di negoziare accordi con Paesi di provenienza e transito in termini chiari soldi per investimenti e cooperazione e assistenza nel controllo delle frontiere contro procedure di rimpatrio facilitate e centri *in loco* per l'accertamento dello *status* di rifugiato e/o di migrante economico. Un lavoro in questo senso, fatto bene, era iniziato in Niger: occorre verificare a che punto siamo. Infine, in questo contesto è purtroppo ineludibile lavorare con la Libia. Gli accordi di cooperazione sono stati siglati da Governi di centrosinistra e centrodestra e voglio dire agli amici di sinistra che è facile chiedere ora di farli saltare, quando non si è al Governo e non si devono affrontare le conseguenze delle aperture di quella rotta. *(Applausi)*. Allo stesso modo la destra non può continuare a ignorare che spesso la Guardia costiera libica è connivente con i trafficanti. Pertanto, bisogna insistere per avere personale Frontex anche sui mezzi della Guardia costiera libica. Il quarto principio prevede di implementare realistiche strategie di redistribuzione e regolarizzazione dei migranti. Sapete che i migranti in Italia sono da dieci anni 450.000, mentre parlavate di invasione? Ma che cosa è successo? Dove sono andati? Sono andati tutti in Europa. Quando parliamo di redistribuzione, dobbiamo considerare che 450.000 migranti sono rimasti; gli altri sono andati in Europa e, se ti metti a litigare con gli altri Paesi europei, rafforzano i controlli alle frontiere e i migranti restano in Italia.

perché ne rimpatriò meno di Alfano e oggi la media è di 5.300 rimpatri contro i 26.000 della Germania, perché non facciamo rimpatri incentivati. Aggiungo, inoltre, perché aprite i flussi - io sono d'accordissimo e non regolarizzate intanto chi trova un lavoro in Italia? Sarebbe una cosa di tutta logica. *(Applausi)*. Il quinto principio riguarda la riorganizzazione delle strutture interne. Abbiamo bisogno di un'agenzia

e altri centri di prima accoglienza, oggi siamo a più dell'80 per cento di saturazione. L'estate così non la affrontiamo. Ultimo punto: lo *ius culturae*. Non dovrei essere io a spiegare a voi, cultori della romanità, che l'allargamento della cittadinanza lo abbiamo inventato noi. Al contrario delle *polis* greche, fondate sullo *ius sanguinis*, dalla sua fondazione Roma ha costruito la propria egemonia sull'Italia e sul mondo allargando il diritto di cittadinanza. Collegare il diritto di cittadinanza al completamento di un ciclo di studi non vuol dire annacquare la nostra identità, signora Presidente, ma forgiare nuovi italiani e dare forza alla Nazione. Onorevole Presidente, di tutto l'inutile rumore prodotto in Italia relativamente a pressoché ogni questione, quello sui migranti è stato il più dannoso e immorale. La destra, quando era all'opposizione, ha usato termini orrendi, ha fatto battute truculente, ha dileggiato i disperati dipingendoli come crocieristi con telefonini e animali domestici; avete parlato di sostituzione etnica e di islamizzazione pilotata. Ora tutto questo rumore è stato spento dalla realtà. Spero non inizi quello di segno opposto. Quello che oggi vi chiediamo è di deporre il rumore di ogni colore e di lavorare insieme per affrontare per tempo quella che descriviamo da dieci anni come un'emergenza, ma che emergenza evidentemente non è. Dobbiamo arrivare in Europa con un piano realistico, circostanziato e rispettoso del diritto internazionale.

Signor Presidente, ci sono occasioni in cui l'Italia deve parlare con una voce sola, occasioni in cui la politica dovrebbe comprendere che, per contare davvero in Europa e avere rispetto e considerazione dall'Europa, il mandato parlamentare dovrebbe essere pieno e convinto. Ebbene, oggi è una di queste occasioni. Siamo alla vigilia di un appuntamento cruciale per le sorti delle politiche che in questi anni sono state al centro del dibattito europeo, a cominciare proprio dall'immigrazione; un vertice al quale dovremmo arrivare tutti con la stessa consapevolezza, ossia che l'Italia non può farcela da sola, ma ha bisogno dell'Europa, così come l'Europa ha bisogno di noi, che rappresentiamo la porta di accesso per entrare nell'Unione. Questa porta d'accesso spesso viene scardinata con violenza da parte dei mercanti di uomini. È quindi quanto mai è necessario che l'impegno per il riconoscimento della cosiddetta dimensione esterna delle frontiere europee, rilevante passo in avanti compiuto grazie al nostro Governo per una nuova politica di cooperazione verso i Paesi di partenza e di transito dei migranti, venga concretizzata concretizzata con adeguati stanziamenti. Allo stesso tempo, non è più rinviabile un piano per una gestione comune delle frontiere esterne e dei rimpatri. Ben venga dunque il piano presentato qualche giorno fa dalla Commissione, che lei ha richiamato e che va finalmente nella direzione richiesta dall'Italia, ribaltando la narrazione dell'accoglienza indiscriminata, tanto cara alla sinistra. Dopo anni di parole al vento e di retorica delle porte aperte, presidente Meloni, aver finalmente posto con fermezza la questione migratoria sui tavoli europei è un grande merito che le va riconosciuto e che va riconosciuto a questo Governo. L'inflessibilità verso l'immigrazione illegale e l'apertura di canali legali attraverso i decreti flussi sono due facce della stessa medaglia, quella di un'immigrazione finalmente gestita e non subita, in cui non siano gli scafisti a decidere chi può entrare e chi no e non siano gli italiani a subire le conseguenze di flussi irregolari che poi si scaricano drammaticamente su tutti noi in termini di lavoro nero, sfruttamento e delinquenza. Me lo lasci dire, Presidente: in una fase così decisiva per l'Italia, chi a sinistra preferisce speculare sulle tragedie, raccontando menzogne e cercando di dare dell'Italia l'immagine di un Paese in cui chi è in difficoltà in mezzo al mare viene lasciato morire, finisce per fare proprio il gioco di quei Governi europei che hanno sempre puntato a fare dell'immigrazione un problema solo dell'Italia e degli altri Stati costieri. E finisce anche per fare il gioco degli ignobili trafficanti di esseri umani, che approfittano di un'Europa divisa per lucrare sulla pelle dei disperati. Chi tifa per il fallimento del prossimo Consiglio europeo, tifa per la sconfitta dell'Italia *(Applausi)* e, ancor peggio, vuole il male dei migranti che a parole sostenete e proteggete. Questa, signori miei, si chiama ipocrisia. Noi non ve lo consentiremo, perché difenderemo l'Italia, il nostro interesse nazionale e la volontà sovrana degli italiani che ci hanno chiesto di fermare l'immigrazione irregolare. Difenderemo il buon nome delle nostre Forze dell'ordine e delle nostre Forze armate, che ogni giorno rischiano la vita anche per salvare vite umane da questo indegno traffico. *(Applausi)*. Lo faremo in ogni sede, in questo Parlamento e nei consessi internazionali, dove finalmente siede un'Italia orgogliosa della propria storia e sicura delle proprie ragioni. Tutto questo è possibile oggi, signor Presidente, grazie finalmente a un Governo politico, che finalmente si pone in Europa con la testa alta e la schiena dritta, non sbattendo sterilmente i pugni sul tavolo, ma affermando con pragmatico buonsenso le solide ragioni del nostro interesse nazionale su tutti i *dossier* e su tutti gli argomenti. Sono fiduciosa che questa postura, finalmente nuova per un Governo italiano, una postura che non vedevamo dai tempi dell'ultimo Governo guidato dal presidente Berlusconi, darà i risultati che tutti quanti speriamo e che saranno certamente utili per il futuro dell'Italia. Lo abbiamo visto anche sulle questioni ambientali, cui il Presidente del Consiglio ha accennato nel suo intervento: ne è un esempio quello che è avvenuto sul regolamento che vieta l'immissione in commercio, a partire dal 2035, delle auto a benzina o diesel, un provvedimento figlio della più becera ideologia ultra-ambientalista, che finirà col desertificare il settore automobilistico e col consegnarci alla Cina, che oggi detiene gran parte delle materie prime necessarie alla nostra transizione ecologica. *(Applausi)*. Il tutto senza che il mondo ne abbia il benché minimo beneficio, il tutto per puntare sul verde, mandando però in rosso l'economia di una Nazione e di un Continente. Allo stesso modo, ci auguriamo che si allarghi il fronte dei Paesi contrari alla direttiva sulle case *green*, perché certamente tutti vogliamo perseguire l'efficientamento energetico dei nostri edifici, ma questo non può essere fatto in così pochi anni, senza incentivi e senza alcuna flessibilità. Su questo il presidente Berlusconi è stato chiarissimo: la casa è il primo investimento delle famiglie, l'80 per cento degli italiani vive in una casa di proprietà, che quasi sempre è stata acquistata grazie ai risparmi di una vita, magari chiedendo prestiti alle banche. Ecco perché per noi la casa è sacra. *(Applausi)*. Non accettiamo che le sinistre europee, con il plauso del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle, provino anche solo a imporre una patrimoniale, neanche tanto mascherata, sui risparmi degli italiani. Mi auguro che al nuovo corso del Governo italiano si possa presto accompagnare un nuovo corso della politica europea, che prenda spunto proprio dall'Italia. Permettetemi, a tal proposito, La maggioranza Ursula, nata per garantire governabilità, ora ha il fiato corto. C'è bisogno di un centrodestra di governo anche a Bruxelles e a Strasburgo, che sappia riportare realismo e pragmatismo: lo dico da Presidente dei senatori di Forza Italia, che rivendica con orgoglio l'appartenenza alla famiglia dei popolari europei, della quale siamo perno insostituibile. La grande coalizione PPE-socialdemocratici è uno schema che non basta più e che oggi non è più in grado di dare le risposte che centinaia di milioni di europei si aspettano. Presidente, mi permetta di notare, con una certa preoccupazione, che la risposta della Banca centrale europea, che ha disposto un ulteriore aumento di mezzo punto dei tassi di interesse, rischia di essere inadeguata, perché - lo diciamo con rispetto dell'autonomia di Francoforte - rischia veramente di minare la risposta europea in questa fase di difficoltà economica, aggravata ancora dalla guerra, che dopo un anno non smette di mietere vittime. La solidarietà con l'Europa, con l'Occidente e con l'Alleanza atlantica è una bussola della nostra politica estera. Per questo di fronte alla crisi ucraina, che da un anno lacera l'Europa e ha riportato gli orrori della guerra nel cuore del nostro Continente, Forza Italia ha sostenuto con coerenza le decisioni del Governo italiano e dei nostri alleati dell'Occidente. A maggior ragione, sosteniamo oggi con assoluta convinzione le sue parole, Presidente, e le scelte che questo Governo farà. Non abbiamo avuto e non abbiamo oggi alcun dubbio, alcuna esitazione nel condannare l'aggressione russa ad uno Stato sovrano. La risposta compatta dell'Occidente non può che essere dunque la risposta dell'Italia. Al tempo stesso sappiamo che la strada per difendere la libertà e la sovranità del popolo ucraino non è in contraddizione con la ricerca di una soluzione politica che ponga fine alla perdita di vite umane e alla sofferenza delle popolazioni. L'Europa, come il presidente Berlusconi chiede da tempo, deve diventare soggetto politico e svolgere un ruolo importante per la pace e la sicurezza di tutti, e prima di tutto del popolo ucraino che va messo in condizione di potersi difendere sempre. Per concludere, Presidente, come è evidente dai numerosi *dossier* sul tavolo, tutti delicati e fondamentali, l'appuntamento del 23 e del 24 a Bruxelles, rappresenta uno snodo fondamentale per il futuro del nostro Paese e per quello dell'Europa tutta. È per questo che siamo orgogliosi e rassicurati dal fatto che ad affrontare questo snodo ci sia finalmente un Governo autorevole che lavora nell'esclusivo interesse dell'Italia e degli italiani. Annuncio pertanto il voto favorevole di Forza Italia

*recovery fund*: «l'Italia esce in piedi; (...) riconosco a Conte di essersi battuto»; 21 luglio 2020. Chi l'ha detto, presidente Meloni? presidente Meloni? L'ha detto lei il 21 luglio 2020 e adesso ci ha appena regalato l'ennesima delle sue piroette, un cambio di posizione rispetto a quanto detto poco tempo fa, soltanto per insultare un suo avversario politico. Ci vuole del fegato, presidente Meloni, per capovolgere completamente la realtà. Ora è lei la Presidente del Consiglio, è a lei che tocca tenere la schiena dritta, come ha fatto il presidente Conte, e andare in Europa per sfidare i Paesi frugali *(Applausi)*, la sua Ungheria e tornare con 209 miliardi. del fegato per stravolgere la realtà, come ha appena fatto lei, di fronte invece a un Presidente del Consiglio che ha avuto il coraggio di dire no al MES quando tutti lo propagandavano come la panacea di tutti i mali.

immeritatamente viene qui a gestire. Riportiamo un minimo di realtà in quest'Aula.

che viviamo un terribile conflitto nel cuore dell'Europa, scatenato da Putin con un'ignobile aggressione ai danni dell'Ucraina. Questo conflitto ha assunto dimensioni sempre più abnormi, quasi fuori controllo, al punto che all'orizzonte si profila nuovamente lo spettro di una catastrofe nucleare. Uno spettro che speravamo tutte e tutti di esserci lasciati alle spalle. Non trova, Presidente, e non trovate, colleghe e colleghi, che sia giunto il momento di fermarsi, di riflettere e chiedersi se quella imboccata sia veramente la strada giusta, se questo sia veramente il modo migliore per aiutare la popolazione civile ucraina. C'è infatti una cosa che fuori da questo Palazzo è chiarissima, ma che a voi non è affatto chiara: la strategia del continuo invio di armi è fallimentare, sta fallendo. mesi assistiamo allo stesso copione; abbiamo iniziato con dispositivi difensivi minimi, poi le munizioni, i missili, i carrarmati. Zelensky vuole ora cacciabombardieri, navi da guerra e sottomarini. Veniamo a sapere addirittura che ci sono militari ucraini sul suolo italiano in addestramento per l'utilizzo dei SAMP/T, il sistema missilistico terra-aria che noi e la Francia ci siamo impegnati a fornire. [**Presidenza del presidente sta facendo crescere ulteriormente la preoccupazione degli italiani. Tanto più alla luce di questo nuovo fatto, ci sono domande a cui non vi potete più sottrarre. L'Italia si sta preparando ad entrare attivamente, con un coinvolgimento diretto, in questo conflitto? Signor Presidente, abbia il coraggio di chiarirlo: stiamo entrando in guerra? Perché se c'è un limite all'*escalation* militare, che vi siete dati, questo limite non è chiaro. Diteci se c'è un limite all'*escalation* militare che vi siete dati! siete dati! Ci vuole onestà intellettuale e questo lo dico anche al Partito Democratico. Chi è per l'*escalation* militare non può essere anche per un percorso diplomatico che porta alla pace. Delle due, l'una: basta ipocrisie, basta portare avanti discorsi contraddittori! *(Applausi)*. alla vostra miopia che l'Italia non può più ambire a giocare un ruolo da mediatore, come era possibile fino a pochi mesi fa. Avete bruciato questa strada, con il vostro furore bellicista, cedendo a Washington ogni decisione che riguarda il conflitto, che però si svolge sul suolo europeo. Presidente Meloni, i cittadini l'hanno votata perché hanno sentito parlare di cose come eurocrazia e pacchia finita in Europa. Devo dire che è francamente imbarazzante vederla oggi affannarsi per cercare di accreditarsi nei salotti buoni, proprio di quei tecnocrati che aveva promesso di combattere. La propaganda si è infranta sulla realtà: dall'immigrazione alle trivelle, dalle accise al superbonus, dal no al tetto al contante all'utilizzo del POS, la vostra lista di piroette, inversioni a U ed incoerenze è infinita. anzi, caro Presidente del Consiglio, siamo sorpresi perché abbiamo sentito dire, poco fa, dalla sua viva voce, che l'obiettivo del Governo è una crescita stabile e duratura, perché solo questa è la garanzia di una diminuzione del debito pubblico. Ma dov'è la crescita di cui parla? Forse lei non lo ricorda, ma all'ultima legge di bilancio ha allegato una previsione di crescita dello 0,6 risultato che peraltro, con la stretta della politica economica della BCE, rischia di essere ancora inferiore e di riportare l'Italia nel funesto limbo tra stagnazione e recessione. Il tutto dopo che il PIL italiano era cresciuto nell'ultimo biennio del 10,7 per cento *(Applausi)*, grazie alle coraggiose politiche espansive che noi abbiamo messo in campo, che il presidente Conte ha messo in campo, contro l'austerità. Come si cresce, tagliando gli investimenti? Che si chiamino superbonus o transizione 4.0, state tagliando tutto, eppure parlate di crescita! ricordi che il debito pubblico, proprio grazie alle nostre politiche espansive, è diminuito di 11 punti, dal 2020 ad oggi. Ormai siamo abituati, Presidente, al fatto che tra le sue parole e i fatti ci sia un abisso, come sull'immigrazione. Mi consenta: *slogan* e propaganda, ma intanto gli sbarchi sono triplicati. I numeri sono questi e sono impietosi La verità è questa, Presidente: altro che patriota! Lei si è fatta dettare la politica economica da Bruxelles e la politica estera da Washington. *(Applausi)*. Non ha nemmeno provato ad incidere nell'interesse della Nazione. Non proprio un atteggiamento da fratello - o da sorella, sempre che non si offenda - d'Italia: non trova? A questo Consiglio europeo non solo l'Italia dovrebbe farsi sentire per evitare un'*escalation* militare e provare a intavolare trattative di pace, ma anche per evitare un pericoloso ritorno al passato, quando cioè alle crisi si rispondeva con tagli alle spese sociali e agli investimenti e con aumenti della pressione fiscale. Il patto di stabilità - lo diciamo chiaramente in quest'Aula - non può essere ripristinato come se nulla fosse, dal 1o gennaio 2024. Purtroppo, invece, cosa state facendo? Con il ministro Crosetto state brigando affinché l'Europa si decida a scorporare quali investimenti dal patto di stabilità? Non quelli *green*, che state ostacolando, non quelli sulla sanità, non quelli sulla scuola che cade a pezzi, ma quelli per le armi. Lei e la sua maggioranza, Presidente, rispondete direttamente alle *lobby* delle armi *(Applausi)*, come dimostra anche l'approvazione del famoso emendamento Foti, inammissibile a norma di Regolamento, che autorizza i cacciatori a sparare anche in città. Mi lasci dire, Presidente, che lei mente

Eravate d'accordo con Draghi per aumentare da subito le spese militari e dare 15 miliardi sull'unghia per raggiungere il 2 per cento dell'accordo NATO. *(Applausi)*. Noi lo abbiamo impedito; noi abbiamo impedito che l'Italia si dissanguasse per le armi.

faccia gli interessi degli italiani a Bruxelles e non torni a mani vuote. Le ho dato del tempo aggiuntivo abbondante *(Commenti)*, non certo per uscire dai canoni della buona educazione.

colleghi senatori e colleghe senatrici, nel comunicare il nostro voto favorevole alla risoluzione di maggioranza - ringraziamo tutti i membri delle Commissioni, della Camera e del Senato, che hanno lavorato alla risoluzione e lo stesso Governo esprimiamo forte preoccupazione per come stanno andando le cose sul fronte della guerra tra Russia e Ucraina. Le iniziative di mediazione di alcuni Paesi vengono subito accantonate e giudicate non credibili ancora prima di essere attentamente analizzate. L'obiettivo della cessazione delle ostilità sembra più una dichiarazione di principio. Anzi, si sente parlare costantemente di offensiva: la Polonia è pronta a inviare addirittura i caccia. Il problema non è il sostegno militare all'Ucraina; il problema è una corsa ad armamenti sempre più potenti, con il rischio di un incidente da cui non si possa più tornare indietro. Siamo certi che una *escalation* del conflitto riuscirà a tenere lontana la guerra dall'Europa e dal nostro Paese? Non esiste una soluzione militare per questo conflitto: né Kiev, né Mosca possono vincere. Queste sono affermazioni del Capo di stato maggiore della Difesa italiana, italiana, esattamente identiche a quelle fatte dal Capo di stato maggiore degli Stati Uniti, così come ci sono esperti analisti americani vicini al dipartimento vicini al dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che invitano alla cautela perché credono molto possibile un'*escalation* e che questa possibilità aumenti esponenzialmente ogni giorno che passa se non si arriva ad una soluzione diplomatica. saggi consigli - verrebbe da dire - davanti ai quali la politica sembra restare sorda. Davvero qualcuno pensa di sconfiggere militarmente la Russia? La storia dovrebbe insegnare qualcosa e chi dimentica la storia è condannato a ripeterla.

In questi tre mesi un po' di equilibrio e un po' di stallo c'è stato, ma purtroppo dobbiamo constatare che ben poco è stato fatto o ben pochi sono stati i passi in avanti sul fronte del cessate il fuoco e anche della tregua; ci siamo trovati di fronte al deserto della diplomazia. Comprendiamo che la Polonia, i Paesi baltici, i Paesi dell'Europa orientale, essendo i maggiormente esposti e anche per la loro storia, facciano valere il loro giusto peso all'interno dell'Alleanza atlantica, a nostro giudizio servirebbe più equilibrio. Occorre recuperare il ruolo storico dell'Italia insieme ai Paesi del Centro Europa per favorire il dialogo e almeno la tregua. Contiamo su di lei, signora Presidente del Consiglio. L'Italia conta su di lei. Sento dire dalla gente che lei è una tosta, non solo perché ha avuto il coraggio di andare all'assemblea della CGIL, ma per tutta una serie di motivazioni. Comprendiamo non sia facile fare delle proposte in ambito di Alleanza atlantica, perché si rischia subito di essere accusati di collaborazionismo e di complicità con il nemico; tuttavia, se è vero che stiamo combattendo la battaglia per difendere la libertà dell'Occidente, dobbiamo essere anche pronti a difenderla all'occorrenza in casa nostra. Che libertà è quella che criminalizza qualsiasi idea che si discosti, anche di un millimetro, dal pensiero dominante? Mi faccia dire che assomiglia più ad una dolce tirannia. Facciamo presente nell'Unione europea che compito dell'Alleanza atlantica dovrebbe essere non solo quello di fornire aiuti all'Ucraina, ma anche quello di fornire aiuti economici per stabilizzare i Paesi del Nord Africa, a partire dallo sblocco degli aiuti alla Tunisia (in questo caso c'è di mezzo anche il Fondo monetario internazionale), proprio evitando partenze di massa ed evitando un'emergenza di carattere umanitario, mettendo in sicurezza il Mediterraneo allargato in virtù di quella che gli esperti chiamano la cosiddetta guerra asimmetrica. Serve rafforzare il fianco Sud, anche l'Italia è un Paese esposto. Serve un piano per l'Africa, per farla prosperare, non può essere sfruttata per le risorse che ha. A proposito di battaglie per la tutela dei diritti, come ha ricordato bene anche lei, va affermato il diritto a non emigrare, a vivere e prosperare nella propria terra di origine. La soluzione non può essere quella di portarli tutti in Italia senza sapere poi come gestirli. Il giornalista Federico Rampini di recente ci ha ricordato che l'immigrazione incontrollata l'hanno sempre voluta i capitalisti; lo scriveva un certo Karl Marx nel 1870 a proposito dell'immigrazione irlandese: così è inevitabile che una massa di immigrati che arrivano favorisca solo manodopera a basso costo. Umberto Bossi lo diceva trent'anni fa, altro che salario minimo. un mondo che va al contrario, come si evince anche dalle direttive europee sul tema della transizione energetica, che tra auto elettriche e case *green* rischia di far pagare il prezzo più alto proprio alle fasce più deboli, di cui si sente tanto parlare di quest'Aula. Sulle auto è facile, basta vedere quanto costano; sulle case *green* basterebbe sentire l'audizione che ha fatto l'Associazione bancaria italiana per rendersi conto dei rischi di stretta sui mutui che ci saranno in futuro favorendo solo chi comprerà abitazioni con classe energetica alta e con il conseguente deprezzamento di chi invece possiede oggi e paga un mutuo su una casa di classe energetica più bassa. Per non parlare dei limiti imposti ad agricoltori e allevatori, accusati di essere fonte di inquinamento solo perché qualcuno a Davos, un *club* privato di non eletti, ha deciso che vuole fare *business* su carne sintetica e insetti. Altro che tutela dell'ambiente: alla base di tutto - non prendiamo in giro i nostri cittadini - ci sono solo gli interessi di qualche potente o di qualche multinazionale. Visti questi presupposti, Presidente, le auguriamo un bel in bocca al lupo al Consiglio europeo; vista la situazione, di sicuro ne ha bisogno. Confidiamo nell'opera del suo Governo e nella sua volontà di difendere gli interessi nazionali, anche se sarà durissima, durissima, perché abbiamo l'impressione che in Europa - ma possiamo dire in tutto l'Occidente - dopo aver perso la fede, si stia perdendo anche la ragione.

sul tema della *governance* economica e sulla gestione dei flussi migratori, c'è un non detto che, a mio avviso, va affrontato se il Governo italiano vuole adempiere la sua missione storica, che è quella di aiutare

il più forte attore internazionale in questo momento, la Cina, sta portando all'ordine internazionale per come l'abbiamo conosciuto. La posta in gioco è proprio lì e questa sfida ha bisogno di una risposta all'altezza. Davvero, come Italia, possiamo pensare di rispondere solo richiamandoci alla retorica della nostra Nazione e degli interessi nazionali o dobbiamo pensare come l'Italia può dare un contributo a una nuova Europa? Questo è il punto fondamentale. Parto da qui, dall'azione diplomatica cinese, che ha conosciuto, rispetto ai tempi più lunghi a cui era abituata, un'accelerazione negli ultimi anni. Il motivo che aveva portato il Gruppo del Partito Democratico a votare in dissenso rispetto all'allora Governo Conte I, in cui il sottosegretario Geraci, leghista, aveva dato il via libera, insieme al Governo di allora, alla via della seta senza avere un previo via libera a livello europeo, è sotto gli occhi di tutti che dobbiamo avere a che fare con la Cina e dobbiamo avere rapporti commerciali, ma davvero possiamo pensare di aderire a un progetto che non è solo commerciale ed economico, ma è il progetto, legittimo dal punto di vista cinese, di rivedere l'ordine internazionale senza averne ragionato con i nostri *partner* europei e aver adottato prima una strategia europea? Ancora oggi, quella di Xi Jinping a Mosca è una visita annunciata per dire che, al di là del messaggio chiaro che oggi Mosca è un *junior partner* rispetto a Pechino, su tutte le grandi crisi internazionali Pechino vuole dire la propria, e non è più l'arma commerciale quella prevalente nella sua diplomazia, ma le affianca anche l'arma militare, quella diplomatica e quella politica. La foto che mi ha colpito ancora di più, la scelta che ci ha colpito ancora di più, non è certo la visita a Mosca, ma la foto scattata in territorio cinese in cui il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, è in mezzo ai consiglieri della sicurezza di Arabia Saudita e Iran. Questo che il blocco dell'Est, egemonizzato dalla Cina, parla e vuole egemonizzare anche il blocco Sud (una volta si sarebbe detto quello dei non allineati). Quella è la grande sfida. Come risponde l'Europa? Come risponde anche nel rapporto con gli Stati Uniti? E qui lo chiediamo a lei, Presidente del Consiglio: qual è il modello che vuole seguire? Quello polacco, di affidarsi alla sicurezza

ma quando c'è da parlare di Stato di diritto, del rispetto dei diritti fondamentali, della libertà di espressione, della libertà di orientamento sessuale, delle libertà politiche, della libertà di stampa, si sente con le mani libere? Penso che dobbiamo stare con l'Europa dei Padri fondatori e questo vuol dire costruire, all'interno dell'Alleanza atlantica, un equilibrio tra il pilastro europeo e quello statunitense e ridefinire gli obiettivi a livello di politica internazionale, laddove giustamente gli Stati Uniti ci chiedono di prendere atto che il baricentro si è spostato nel Pacifico, dove risiedono le principali sfide alla sicurezza globale. Nel momento però in cui ci chiedono un investimento in quel teatro geo-strategico, noi dobbiamo chiedere loro una mano

o a quale modello di democrazia ispirarsi, ma solo ed esclusivamente i cittadini ucraini. *(Applausi)*. Loro si stanno battendo per questo principio e noi siamo al loro fianco per questo motivo. È l'idea di *soft power* europea che in qualche modo ci distingue e fa sì che ci battiamo per quei diritti, per quei principi, per quei valori e per quelle libertà in Europa e contestiamo la Polonia e l'Ungheria, quando si oppongono alla difesa di quei diritti. Lo facciamo in Europa e lo dobbiamo fare ad ogni latitudine. Per questo motivo, Presidente, le chiediamo un intervento forte all'interno di questo Consiglio europeo quando si affrontano i temi della politica estera, in modo tale che in tutte le sedi si prenda posizione netta a tutela delle donne e del popolo iraniano che si stanno battendo contro il regime liberticida

un segnale molto forte che darebbe anche l'Italia insieme al Parlamento europeo, a fianco degli iraniani che protestano in questo momento. *(Applausi)*. Se scegliamo il modello dei Padri fondatori, quello del mutuo soccorso, della solidarietà, della responsabilità comune

a quella dall'elettrico cinese. È una battuta fin troppo facile: sappiamo che è tutto maledettamente più complesso; non invidiamo il ministro Fitto per il lavoro che deve svolgere in Europa; sappiamo qual è la complessità dei negoziati e anche la capacità di costruire spesso alleanze a geometria variabile per trovare soluzioni.

Material Act, perché sappiamo che le materie prime fondamentali per affrontare la transizione ecologica e digitale sono in altri Paesi e abbiamo bisogno di recuperarle. lei, perché adesso è lei il Presidente del Consiglio e non è più all'opposizione - quali sono le politiche industriali che vuole affiancare a questi grandi progetti europei, per far sì che non rimaniamo ostaggio delle contraddizioni anche di questo impetuoso cambiamento. Da ultimo, c'è il delicato tema dei flussi migratori. Da una Presidente del Consiglio ci attendiamo risposte all'altezza delle sfide che abbiamo davanti, per cui abbiamo trovato fuori luogo le parole che ha rivolto nei confronti della nostra collega Tatiana Rojc.

che abbiamo scolpiti nella nostra Carta europea dei diritti e nelle nostre Costituzioni: al centro ci sono la persona umana e l'altissimo valore attribuito alla vita umana. Le leggi del mare

Non ci rassegniamo all'idea che in un tribunale italiano i trafficanti che speculano sulle tragedie delle persone e li condannano a morte si trovino insieme a chi, invece, rischia in proprio per salvare quelle vite. Noi vogliamo affrontare questo nuovo approccio difficile e complicato. La lettera della von der Leyen apre una prospettiva interessante, quella dei corridoi umanitari (480 milioni per farli), dei ricollocamenti su base obbligatoria e di far pagare quei Paesi che in passato non hanno voluto prendersi neppure un rifugiato e lo vogliamo fare con uno spirito che non mette in campo solo strumenti economici.

che abbiamo bisogno anche di iniziative politico-culturali, perché sono l'antidoto migliore alle tentazioni neopolitico-imperialiste. Noi siamo l'Europa, abbiamo una storia diversa: differenziamoci.

abbiamo una certezza sul prossimo Consiglio europeo e questa certezza è che l'Italia vi andrà da protagonista e non da comprimaria. Chi ci rappresenterà, presidente Meloni, non andrà alla ricerca di *photo opportunity* o di pacche sulle spalle da parte dei presunti *leader* che contano, perché sarà un *leader* che conta perché rappresenta l'Italia, Stato fondatore dell'Unione europea, terza economia oggi in Europa e tra le prime 10 Ci sarà poi anche qualcosa di più degli ultimi mesi: conterà perché ha l'appoggio di una coalizione coesa, ha una prospettiva di di lungo periodo e non i soliti nove-quindici mesi che abbiamo quasi sempre visto in passato ed è espressione diretta del voto degli italiani, cosa che è apprezzata nei Paesi democratici. ancora di più perché conosciamo bene la sua determinazione e la preparazione accurata con la quale arriva a tutti gli incontri, cosa che le ha fatto guadagnare, insieme al sostegno di cui gode, il rispetto e il prestigio internazionali anche in questi pochi mesi. Sulla questione dei migranti, ha già spiegato accuratamente la posizione:

al controllo della legge e non dei trafficanti di esseri umani. Questo è molto chiaro e la politica del Governo in ciò è stata lineare e coerente.

le dichiarazioni del presidente del gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, Iratxe García Pérez, che ha detto che il nostro Presidente del Consiglio ha le mani sporche di sangue,

sarebbe stata informata che, negli anni dal 2014 al 2017, con Presidenti del Consiglio del Partito Democratico, i morti nelle acque intorno all'Italia sono stati 13.700. *(Applausi)*. che non sia stato un esponente del Partito Democratico a informare la capogruppo spagnola del gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo.

coraggiosamente ipotizzato e chiamato "piano Mattei", cioè un piano nei confronti dell'Africa che supplisca a decenni di assenza da parte dell'Unione europea, anche perché negli ultimi negli ultimi dieci anni sembrava, a livello internazionale, che l'Unione europea partisse a nord delle Alpi. A sud delle Alpi non c'era nulla e dunque perché interessarsi dell'Africa? l'Africa è un versante importantissimo per l'intera Europa e naturalmente per l'Italia, che è la Nazione più vicina all'Africa. Con lei, presidente Meloni, l'Italia ha una posizione ben chiara sulla questione ucraina e nel supporto all'Ucraina, cosa che non si può dire, evidentemente, dell'attuale opposizione. Faccio presente che il partito Alleanza Verdi e Sinistra, alleato principale del Partito Democratico nelle elezioni di pochi mesi fa, ha scritto nella sua risoluzione di voler interrompere completamente qualsiasi supporto di carattere militare. La stessa cosa è scritta nella risoluzione del MoVimento 5 Stelle,

con dati estremamente positivi. Contrariamente alle previsioni dei catastrofisti di casa nostra, le cose sono andate all'opposto. Altro che tracollo: la borsa è salita del 26 per cento dalle scorse elezioni, lo *spread* è sceso di 37 punti, il prezzo del gas, da quando si è insediato il Governo, è sceso del 58 per cento, non certo solo per l'azione italiana, ma anche grazie all'azione dell'Italia a livello internazionale. Addirittura il debito è sceso di 15 miliardi. Ho sentito poc'anzi la collega dire che il debito pubblico negli scorsi due anni sarebbe sceso dell'11 per cento, forse facendo qualche acrobazia con la percentuale sul PIL, basandosi sul fatto che nel 2020 il

2021 a ottobre 2022, il debito pubblico è aumentato di 199 miliardi: questi sono i dati della Banca d'Italia. Il nostro Governo difenderà gli interessi degli italiani e condivide gli obiettivi di difendere l'ambiente (chi è più attaccato alla difesa dell'ambiente dei conservatori?), ma bisogna farlo in modo razionale, possibile e socialmente ed economicamente sostenibile. Rispetto alla direttiva sulle case*green*, rivendichiamo con orgoglio di esserci opposti, sia come Governo, sia come Gruppi parlamentari di tutto il centrodestra al Parlamento europeo. Tante volte avete parlato, anche adesso, del carovita che è aumentato e dell'inflazione, che non è un fenomeno che si è verificato solo da ottobre scorso, quando si è insediato il nuovo Governo, ma era già ampiamente presente nei mesi precedenti.

non meno di 45.000 euro, salvo ulteriori aumenti dovuti all'accumularsi in tutta l'Europa di persone che userebbero le stesse materie prime e gli stessi materiali, magari anche le stesse imprese; 45.000 euro che graverebbero su ogni proprietario di unità abitativa e che per gli inquilini, che ovviamente non li sosterrebbero direttamente, rappresenterebbe (basta fare alcuni semplici calcoli) un aumento dell'affitto di non meno di 200 euro al mese. *(Applausi)*. Se questo è un modo per aiutare i cittadini di fronte all'aumento del costo della vita, direi che è il modo sbagliato.

farebbero perdere centinaia di migliaia di posti di lavoro e moltissime persone dovrebbero rinunciare ad avere l'auto. Ricordo una cosa: il senatore Misiani ha detto che l'alternativa dell'elettrico è irrinunciabile ed importantissima; anche noi siamo d'accordo che è importantissima, ma allora come mai negli scorsi anni nessuno ha pensato di fare anche solo un impianto per lo smaltimento delle batterie al litio? Le auto elettriche hanno le batterie, che alla fine devono essere in qualche modo smaltite e in Italia non c'è neppure un impianto. Penseremo anche a questo, ma non è facile riuscire a fare tutto subito. Lo faremo, una prospettiva davanti. Presidente Meloni, lei va al Consiglio europeo di Bruxelles con il sostegno convinto della maggioranza del Parlamento

che tra poco più di un anno si voterà per il Parlamento europeo e l'Italia potrà avere ancora più forza.

10, 12, 14, 15 e 16 delle premesse e dei punti 6 e 7 del dispositivo, con la riformulazione del punto 10,

La seduta è sospesa. Gentili senatrici e senatori, lo scorso 3 marzo, come sapete, pochi giorni prima che compisse sessant'anni, ci ha tragicamente lasciato il senatore Bruno Astorre. È un evento che ha scosso l'opinione pubblica e che ha lasciato un vuoto incolmabile non solo per i suoi familiari e i suoi amici, ma in tutti noi, in tutti coloro che lo hanno conosciuto, frequentato o che hanno avuto semplicemente il piacere e l'onore di condividere con lui un tratto della vita istituzionale della Nazione. Egli è stato consigliere comunale, provinciale e regionale; è stato assessore regionale del Lazio e nel 2013 è diventato senatore della Repubblica. Astorre si è sempre distinto per competenza, educazione e come mi hanno confermato anche gli esponenti di forze politiche diverse dalla sua, a partire dal ministro Lollobrigida, che ha tenuto ad essere oggi presente, in quanto lo ha sempre conosciuto da vicino. Democratico cristiano popolare fino a diventare il coordinatore regionale del Partito Democratico, ha saputo incarnare la politica dei nostri giorni mantenendo salde le tradizioni, a partire dal radicamento territoriale e l'attenzione ad elettori e cittadini. La sua scomparsa è un dolore per tutti noi. Lo abbiamo salutato nella camera ardente, che il Senato ha voluto si tenesse nella sala Nassirya, a partire da chi, come i colleghi del Partito Democratico, lo ha frequentato anche fuori da quest'Aula più di molti di noi.

Colleghi, vi invito a osservare un minuto di raccoglimento in memoria del senatore Bruno Astorre.

Era il più allegro e il più cordiale tra di noi: era colui che ogni mattina abbracciava chi incontrava, fuori da quest'Aula e in quest'Aula, con un sorriso; un abbraccio restituito, enorme, imponente,

con l'amore, la dolcezza e la forza incredibile delle parole di Francesca; con il dolore composto e silenzioso di Francesco; con quella fila - fatemelo dire - struggente di decine e decine di sindaci, di qualsiasi colore politico, con i fuochi d'artificio sparati alla fine della cerimonia nel cielo dei suoi colli; una cosa strana alla fine di una cerimonia religiosa, quei fuochi d'artificio sparati nel cielo dei suoi Castelli come ultimo saluto. alla domanda su chi è stato Bruno Astorre era tutta nell'abbraccio di quel campo sportivo: un uomo che si è fatto voler bene da tutti perché ha fatto della politica uno strumento per fare del bene alle persone, non soltanto attraverso gli atti legislativi, che riguardano la generalità delle persone - come pure è giusto fare - ma del bene fatto alle singole persone, impegnandosi per risolvere ogni problema, per aiutare in ogni difficoltà. Nella camera ardente sono stato qualche tempo di fianco a Francesca ed era emozionante vedere in quella fila degli sconosciuti che si presentavano dicendo: Bruno Astorre mi ha aiutato in un momento di difficoltà; mi ha risolto un problema; mi ha cambiato la vita; lo ringrazio perché mi ha aiutato quando avevo bisogno. Può sembrare un metodo forse un po' antico, apparentemente, ma autentico, di gestire il rapporto con gli elettori. Lo ha imparato da ragazzo nella Democrazia Cristiana, quando si riteneva allievo di Severino Lavagnini, un altro senatore importante in quella zona della provincia di Roma, quando la politica in tutti i partiti era davvero popolare ed era fatta di contatto, di ascolto. I *post* e i *tweet* non sostituiranno mai la verità di una stretta di mano, di una pacca sulle spalle, di uno sguardo diritto negli occhi. Bruno voleva le preferenze: quante discussioni. Voleva che nella legge elettorale tornassero le preferenze. Ne aveva parlato con molti di voi. Io e lui abbiamo avuto molte discussioni, perché io ne sollevavo i rischi e lui mi sottolineava i pregi del contatto diretto con le persone. Astorre era un politico preparato, raffinato, dietro quella ricerca voluta di semplicità. la laurea in economia con 110 e lode alla LUISS. Lo ha ricordato il Presidente: amministratore locale; assessore regionale ai lavori pubblici, perché voleva occuparsi delle strade, di cose concrete; Presidente del Consiglio regionale; segretario regionale del Partito Democratico; e poi, e soprattutto, senatore, l'orgoglio di essere senatore. Una volta, in una delle ultime tornate elettorali, gli proposi di candidarsi alla Camera e lui mi guardò malissimo dicendo: io sono senatore e voglio restare al Senato, che è la mia casa. Dovremmo anche interrogarci su cosa abbia voluto dire con "chiudere qui col suo percorso terreno", chiuderlo al Senato. Cosa ci ha voluto dire? E poi la lezione di volerci bene tra avversari: in Bruno gli avversari riconoscevano la verità, la passione, le stesse cose che lui sapeva riconoscere in molti degli avversari. E quando le riconosceva diventava amico, nonostante lo scontro restasse e diventasse magari ancora più duro. È una lezione per tutti noi: non soltanto recuperare, come sarebbe giusto, il rispetto degli avversari; non soltanto evitare inutili cattiverie, ma qualcosa di più, che in quest'Aula sia di esempio per tutti, ossia riconoscere che anche nell'avversario più lontano, con le idee più diverse, più contrapposte, più inconciliabili, brucia la stessa passione, freme lo stesso amore per la politica come strumento per migliorare il mondo e migliorare la vita delle persone.

il sindaco coprì i muri della città - e solo un sindaco come Giorgio La Pira poteva farlo - con un manifesto del Comune su cui era scritto soltanto: «Da quel chicco di frumento nasceranno tante spighe di grano nuovo». Bruno Astorre è stato un chicco di frumento seminato nella sua terra e da quel chicco di frumento stanno già nascendo tante spighe di grano nuovo.

Ovviamente, non essendo senatore, non lo potevo sapere, ma sono orgoglioso e contento di poter trasmettere le più sentite condoglianze alla famiglia, alla moglie Francesca, ai colleghi senatori e alla comunità politica del PD in particolare, che hanno avuto la possibilità di conoscere e frequentare Bruno Astorre. Certamente nella descrizione del collega Franceschini si è già raccontato quello che valeva: era una persona con la quale si poteva lavorare, si potevano approfondire i temi; si potevano anche, con grande forza e grande convincimento, difendere le idee spesso inconciliabili, ma sempre sostenute con lealtà e rispetto reciproco. Credo che questo sia un esempio di buona politica e lo è stato per tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo. Chi ha lavorato con lui sa quanto fosse pesante la sua presenza, io credo che ancor di più sia pesante la sua assenza. Per chi lo ha conosciuto sul territorio e ha avuto la possibilità di collaborare senza mai fare compromessi; per chi lo ha incontrato negli angoli più sperduti del territorio; per chi ha - come il senatore Franceschini ricordava - la politica come passione fin da ragazzino, avere avversari con i quali poter condividere un percorso da posizioni diverse è emblematico del valore della democrazia, della capacità di rappresentare l'intero specchio di coloro che guardano a noi sperando di vedere in noi persone che risolvono i problemi. Di problemi Bruno ne ha risolti tanti e non in termini clientelari. Il senatore Astorre è arrivato a un livello importante in politica. Abbiamo condiviso i banchi della Provincia di Roma e poi della Regione Lazio in ruoli invertiti, in maggioranza e in opposizione, ma abbiamo sempre trovato il modo di dividere il contrasto politico dalle ragioni che ci univano nella vocazione a dover sempre difendere l'interesse del territorio dal quale provenivamo e nel quale ci eravamo formati. Ho visto a Colonna plasticamente quello che già sapevo: tante persone che intorno a lui sono state quando aveva un ruolo per poter rispondere alle loro esigenze individuali, alle loro rappresentanze come amministratori, e che c'erano in quel giorno per salutarlo, quando per loro

non solo l'opera che Bruno ha compiuto da amministratore e da rappresentante del popolo, ma anche il suo esempio di cordialità, di buona politica e di lealtà. Credo che al di là di tutto mancherà a tutte le forze politiche, a prescindere dalle dalle scelte di carattere individuale, dal senso di appartenenza ai singoli Gruppi. Come ho detto al senatore Franceschini, non sono sicuro di poter restare perché commemorerò Bruno nel mio paese,

ad accendere anche per lui la fiaccola, raccontando ai miei concittadini - molti dei quali lo conoscevano, perché era ultra presente in ogni territorio della provincia di Roma

attraverso un gesto materiale nei palazzi delle istituzioni, in cui magari dedicargli un luogo che possa rammentarne il percorso politico, la volontà e i valori che ha rappresentato, nel nome di un senso di unità che deve sempre più contraddistinguere il nostro modello democratico.

Tante volte ci siamo incontrati, tante volte ci siamo scontrati, tante volte abbiamo discusso, ma soprattutto tante volte abbiamo riso:

pur da ottiche diverse, di saper collaborare per la crescita di un territorio, una persona che amava veramente la politica, quella con la P maiuscola. Aveva una grande capacità di coinvolgimento delle persone, che era il suo grande pregio, la sua grande caratteristica.

per quella voglia di darsi agli altri. Una cosa è importante: Bruno ha dato tanto, ha dato tanto agli altri, ha dato tanto in termini di progettualità politica, ma ha dato tanto agli altri anche in termini di di affetto, di amore, di voglia di risolvere i problemi più banali e più semplici delle persone. È una caratteristica fondamentale per chi ha nel cuore la politica e per chi ha voglia di fare politica. Risulta per ognuno di noi probabilmente incomprensibile il suo gesto. Non siamo riusciti a cogliere l'eventuale disagio che Bruno

ogni giorno, entrando qui, e portava comunque l'allegria. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare in Commissione in questi mesi e comunque, al di là del suo contributo di carattere politico, portava sempre un contributo di giovialità, di allegria, di simpatia e di voglia di fare, mai creare steccati tra le varie posizioni di carattere politico. Questo era il suo grande merito, la sua grande caratteristica. Aveva un profondissimo amore per il suo territorio, che condividevamo. E proprio in virtù del suo insegnamento, spero di poter dare una piccola parte di quello che lui ha dato al nostro territorio, che ci ha accumulato in questa esperienza politica. Ciao Bruno. senatore De Cristofaro spesso la politica, soprattutto a sinistra, si rimprovera e si esorta a cambiare con una formula che è diventata ormai anche un po' un luogo comune: bisogna tornare ai territori e ripartire da lì, si dice molto spesso. che nessuno mai abbia potuto rivolgere quel rimprovero a Bruno Astorre. Non ha mai avuto bisogno di tornare ai territori, perché dall'inizio del suo percorso politico, alla fine degli anni Ottanta la Democrazia Cristiana, dai territori Bruno Astorre non si è mai allontanato. È stato ricordato dal senatore Franceschini, dal ministro Lollobrigida e dagli altri interventi: all'ultimo saluto a Bruno, assieme alle migliaia di persone che lo conoscevano e che gli volevano bene, hanno voluto presenziare e partecipare decine e decine di sindaci del Lazio, anche di diversi schieramenti. Credo che questo dica moltissimo su quale modello di politica ispirasse Bruno Astorre: la consapevolezza che politica vuol dire rappresentare la popolazione e che, per rappresentare la popolazione, bisogna conoscere. Bruno Astorre conosceva il territorio nel quale ha fatto politica per tutta la vita, il Lazio, ed era consapevole di quali fossero gli interessi dei suoi abitanti e degli elettori. Non dimenticava mai che il suo compito e il suo dovere, anche da senatore della Repubblica, erano quelli di rappresentarli al meglio. Per questo si poteva anche non essere d'accordo con lui; ci si poteva anche scontrare - qualche volta è capitato - con il suo carattere forte e determinato, ma non lo si poteva non ascoltare, perché dava voce a interessi, esigenze e domande reali dei cittadini che era chiamato a rappresentare. Quei legami saldissimi con la base, con gli elettori tutti e non solo con i propri, Astorre li ha saputi mantenere anche da senatore, coniugando rappresentanza territoriale e rappresentanza nazionale, come dovrebbe saper fare ogni parlamentare. Ci sono delle vie - tante, come sappiamo - per approdare alla rappresentanza politica. Eppure, io sono convinto che quella seguita da Bruno Astorre sia la via maestra: partire dal basso, che però è soltanto un presunto basso, un basso apparente, cioè dalle amministrazioni locali, e poi conquistare il consenso in virtù dell'affidabilità, della serietà e della conoscenza diretta dei problemi delle persone in carne e ossa e non in virtù, magari, di una smagliante ma superficiale immagine. È esattamente quello, Presidente, che si usava fare nei partiti di massa. Qualcosa di quella lezione, che è anche la lezione di Bruno Astorre, dovremmo saper recuperare tutti, pure in un'epoca così diversa, se vogliamo che la politica torni a essere qualcosa che tocca e coinvolge le masse; se vogliamo, cioè, che la democrazia viva nella sostanza e non soltanto nella forma. Ecco, questa per me è la lezione di Bruno Astorre e credo che dovremmo ricordarla tutti sempre. grazie. Signor Presidente, mi sembra surreale essere qui a commentare la morte di Bruno. Per me era un amico, al di là della politica. Abbiamo passato giornate e serate insieme; siamo partiti insieme nella Democrazia Cristiana, lui nella linea sbardelliana, io nella linea della sinistra DC, poi ci siamo invertiti i ruoli. Bruno Astorre era un vero amico, un avversario politico, ma non un nemico. Pur facendo politica da sponde opposte, ci legavano un rispetto reciproco, una stima profonda e una sincera amicizia. Non poteva avere nemici Bruno, perché era una persona buona e aveva un carattere tranquillo. Lo ha colpito quel male terribile che si chiama depressione, un male ereditario purtroppo, con cui ha convissuto e combattuto a lungo. Questo è il primo insegnamento che ci lascia: si tratta di una patologia vera e propria, che va identificata e curata come ognuna delle gravi malattie che possono colpirci. Sono 2,8 milioni le persone che ne soffrono in Italia, circa 4.000 coloro che, malate di depressione, arrivano al gesto estremo. Noi siamo parlamentari e, come tali, dobbiamo porre al centro della nostra azione politica degli interventi nel Servizio sanitario nazionale anche sul tema della malattia della depressione. Dobbiamo fare ogni cosa per tentare di salvare altre vite, proprio perché oggi sappiamo che la persona che frequentiamo ogni giorno potrebbe decidere domani di non essere più con noi. Il secondo insegnamento che ci lascia Bruno è quello politico. Io che, come lui, sono senatore e responsabile politico nel Lazio, ho vissuto quando era amato e stimato. Faceva politica sul territorio che amava e che a lui deve molto. Le comunità del Lazio devono molto alle sue idee e alle sue soluzioni politiche: si confrontava con tutti, guardandoli in faccia, e per ogni problema era in grado di trovare una soluzione nell'interesse comune, cercando di dare risposte concrete ai problemi reali della gente. Che fosse molto amato nei suoi territori lo sapevamo: lo ha dimostrato anche il fatto che - lo ricordava il Ministro - la celebrazione del suo funerale si è tenuto in un campo sportivo gremito di gente, con manifesti e striscioni. Tantissima era infatti la gente che ha voluto rendergli l'ultimo saluto nella sua Colonna. È grande la passione che metteva nel fare politica e che ha trasmesso a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e frequentarlo. Oggi, quindi, gli siamo debitori, gli dobbiamo tanto amore e gli rendiamo un commosso omaggio, salutando sua moglie Francesca, la sua famiglia e la sua comunità politica. Ciao Bruno, ricorderemo per sempre le tue coinvolgenti battute e il tuo magnifico, indimenticabile sorriso.

il Gruppo per le Autonomie si stringe alla famiglia, ai colleghi, ai dipendenti del PD e a tutti quelli che in questo Palazzo piangono la scomparsa di Bruno Astorre. In questi miei primi mesi al Senato non ho avuto l'occasione di conoscerlo personalmente e di apprezzare direttamente le qualità politiche umane che tanti prima d'ora hanno ricordato nei loro interventi e nelle dichiarazioni pubbliche. Perciò, questo mio breve intervento sarà l'occasione per una riflessione sulla vita del politico. Nell'immaginario sociale, il politico è associato alla forza, al coraggio e all'ambizione, a una persona di potere che viene immaginata con il pieno controllo di sé, un dominio delle proprie emozioni e del proprio io più profondo; una persona di potere che non si ammala e, se si ammala, è in grado anche di gestire la malattia, di camuffarla e superarla. Invece no, noi siamo persone come tutte le altre e ciascuno di noi porta in sé una storia unica e particolare, fatta di forza ma anche di fragilità, di speranza ma anche di paura, di appagamento ma anche di insoddisfazione. Allora, ritengo che questa sia l'occasione per riflettere sulla qualità delle nostre relazioni; su come noi, concentrati sullo scontro politico, possiamo talvolta non comprendere quello che succede a chi ci sta accanto in questa stessa Aula. Questo impoverimento umano, purtroppo, finisce per diventare un impoverimento anche politico. Nel mondo due Capi di Governo donne si sono dimesse per riprendere in mano la propria vita, quasi denunciando un'inconciliabilità tra impegno pubblico e dimensione privata; evidenziando, ancora una volta, come il ruolo politico non sia in grado di coprire le umani fragilità ed, anzi, finisca in verità per disvelarle inesorabilmente. allora che la scomparsa del senatore Bruno Astorre ci sia da monito e ci aiuti a recuperare una dimensione più umana nel nostro fare politica, una maggiore cura nelle relazioni, per non dimenticare mai che, oltre che ciò che rappresentiamo e gli incarichi che ricopriamo, siamo persone come tutte le altre. Buon viaggio, caro collega Astorre, e ancora un abbraccio affettuoso a tutti i suoi cari. Signor Presidente, Bruno Astorre era Bruno Astorre; detta così, può sembrare una frase banale o una ripetizione. Per me è un complimento, perché il collega Bruno Astorre era un grandissimo professionista della politica e tutti noi dovremmo imparare, per le cose che ha detto Dario Franceschini e tutti coloro che si sono succeduti, ad avere quella dimensione della politica. Il collega Bruno Astorre, in tempi di politica liquida, era una solida garanzia; sapevi con chi avevi a che fare quando parlavi con lui. Questo non è facile in un momento come quello in cui noi stiamo vivendo. A me piace ricordarlo come una persona vera che ti trattava allo stesso modo. Capita a chi ha avuto tanto potere e poi lo ha perso tutto insieme di vedere in tante persone un atteggiamento diverso; quando sei potente, tutti ti danno ragione sempre; quando non conti nulla, non ti considerano nemmeno, anche in modo un po' ipocrita. Bruno era uno che quando eravamo all'apice attaccava dei bottoni pazzeschi, lamentando e attaccandoti in modo molto umano, come sapeva fare lui, ad esempio - come ricordava il senatore Franceschini - sulle preferenze. Ricordo una discussione qui, in quest'Aula, su questo tema, in cui provavo, con un po' di *savoir-faire* e di malizia, di dirgli di parlarne con Franceschini, il suo capocorrente, o con Zanda, il suo Capogruppo, un'altra persona cui Bruno era straordinariamente legato. E lui aveva la franchezza di dirti le cose in faccia. Quando invece, viceversa, io ho perso tutto il potere che avevo, Bruno mi guardava con lo stesso carico di umanità e si preoccupava di come stavano i genitori, di come andavano le vicende; aveva un elemento di dimensione umana che non è facile da mantenere. Per questo dico che sapevi con chi avevi a che fare. non ci nascondiamo dietro un dito: non abbiamo saputo fino in fondo con chi avevamo a che fare sotto il profilo umano e personale. È un dolore che ci portiamo dietro tutti. Tutti noi ci domandiamo che forse avremmo potuto, forse avremmo dovuto. Immagino il dolore della famiglia, a cui vorrei davvero mandare un abbraccio doppio; il dolore dei colleghi del PD, di tutti noi. Ci domanderemo sempre se forse non abbiamo sbagliato qualcosa. Sicuramente quella cicatrice non si rimarginerà mai. Penso però che l'unica cosa che possiamo fare in questo momento, credenti e non, è affidarlo per noi credenti a quel Dio di misericordia che vorrei citare con le parole di un laico per rispettare questo luogo. Fabrizio De Andrè quando parla dei suicidi, scrive una canzone che è una delle più belle, immaginando di chiedere al Dio di misericordia di lasciare fiorito il sentiero «Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte ai suicidi dirà baciandoli alla fronte venite in paradiso là dove vado anch'io». E chiede al Dio di misericordia, lui che era laico, «Ascolta la sua voce che ormai canta nel vento. Dio di misericordia vedrai, sarai contento». Può sembrare una strana contraddizione legare la laicità al senso spirituale, ma non c'è alcun motivo per noi che vedevamo quel suo sorriso di poterci dare una ragione per quello che è successo. lo affidiamo, sì, a quel Dio di misericordia, laici e credenti. Ma lo affidiamo soprattutto al ricordo di ciascuno di noi in questo momento perché quel suo sorriso, lui che sorrideva e sapeva sorridere, possa continuare. prendiamo spunto dalla sua capacità di essere una persona vera, un uomo con la u maiuscola, di guardare le persone potenti e meno potenti con lo stesso sguardo di verità. Facciamo anche uno sforzo per guardarci tra di noi, con più rispetto. Forse noi, che non abbiamo saputo capire il male di vivere che Bruno aveva incontrato, potremo fare un tentativo di compassione rispetto a ciò che è accaduto, facendoci carico di avere rapporti diversi tra di noi. Forse anche questo è uno dei grandi messaggi che Bruno Astorre ci lascia: ci lascia: vedere gli altri come persone a cui andare sempre incontro senza pregiudizio. Bruno Astorre era Bruno Astorre: in tempi di camaleontismo della politica, avere a che fare con una persona così per me è stato un motivo di grande orgoglio. Oggi gli vorrei dire semplicemente grazie.

rappresentare parole di cordoglio e di vicinanza ai familiari e agli amici di Bruno. E voglio

È stato detto della passione con cui Bruno, il senatore Astorre, ha fatto politica in questa Assemblea e nelle Commissioni, ma prima ancora nei territori. La sua era una passione genuina, con cui spesso ci si scontrava, con cui si poteva pure litigare. Ma quella stessa passione e quel sorriso poi consentivano anche di fare pace immediatamente, magari di andare a mangiare qualcosa assieme dopo la Commissione, di confrontarci e continuare il dibattito politico che avevamo fatto prima in qualche aula, con la stessa passione, ma con il riconoscimento reciproco della genuinità genuinità con cui si stava cercando magari di risolvere un problema per i cittadini. Ricordo i primi mesi della scorsa legislatura, quando ero Capogruppo di una forza di maggioranza e Bruno era in Commissione, come esponente importante di una forza di opposizione. Mi colpì tantissimo, in quei mesi, il suo avvicinarmi spesso per darmi un consiglio su qualcosa che magari non avevo fatto in modo adeguato, in Commissione o in Assemblea, magari per un intervento che poteva essere declinato in un altro modo. modo. Credo che ci vogliano uno spessore, un'integrità morale e rispetto per la cosa pubblica nel non approfittare magari di una ingenuità o dell'inesperienza politica di un avversario, per dargli invece un consiglio. Questo è un ricordo che porterò sempre nel mio cuore. Ho sentito le parole di Dario, quando ha parlato di frustrazione e della difficoltà nel chiedersi cosa abbiamo sottovalutato, cosa non abbiamo capito e anche Matteo ha detto sostanzialmente le stesse cose. Mi permetto di intervenire, con grande umiltà e sommessamente, dopo averne parlato con Alberto Airola, che ha dedicato a Bruno un saluto in quei giorni e che ha potuto farlo soltanto grazie a un caso e ad un'intuizione di sua sorella, perché Alberto è con noi soltanto per questo motivo. Alberto ha scritto: «Comprendo il dolore e la depressione che possono portare un essere umano ad un atto anticonservativo, è un percorso di dolore insanabile (...). Se posso dire una cosa è che nessuno, nessuno può sapere quello che accadrà, «so che non è di alcun sollievo ma forse può mitigare i sensi di colpa di chi gli è stato accanto». Non voglio aggiungere altro se non dire che, al di là dei sensi di colpa o di quello che ha detto Alberto, Bruno ci mancherà tanto

qui presenti nella giornata di oggi e di tutto il Partito Democratico. Come Gruppo preferiremmo ricordarlo con le parole del senatore Claudio Durigon, che è Sottosegretario, sempre che poi possa intervenire, ai sensi del nostro Regolamento.

possibile soluzione, perché per lui era importante innanzitutto il bene del suo territorio, la provincia di Roma, che lui amava in maniera quasi ossessiva. Era coordinatore regionale del Partito Democratico ed è stato assessore regionale, ma per Bruno Astorre la provincia di Roma era quasi una missione. Conosceva ogni Comune, ogni amministratore dei 120 Comuni che compongono la provincia di Roma; era stimato da tutti,

suo carattere, che era sicuramente pieno di amore; come è stato detto, non lesinava mai a nessuno dei consigli, anche se si era avversari politici. Spesso, soprattutto nei Comuni con meno di 15.000 abitanti, siamo stati anche attaccati, perché la ricerca di soluzioni per i territori veniva scambiata per miseri accordi politici, ma non era assolutamente così perché si è stati sempre avversari, sempre leali. Pertanto Bruno mancherà come punto di riferimento, come persona capace di tradurre la politica in qualcosa di importante, cosa che spesso è mancata. Forse quello che è stato detto è vero. Ricordo che Bruno, forse un mesetto fa, aveva perso il sorriso: stava solo a fumare nella stanza dei fumatori. Io lo vedevo, ma non gli ho dato peso, perché si corre sempre, si pensa sempre

particolari. Io lo vedevo fumare lì e non ho dato peso alla cosa. Questo ti fa pensare che spesso e volentieri, come è stato detto, si è avversari politici ma si vive qui dentro tutti insieme e forse bisognerebbe maggiormente

però ci lascia anche la forza di quello che ci ha insegnato, ossia di essere sempre onesti, perché Bruno, prima di tutto, era una brava persona.

della nuova situazione nella Regione e di come fosse disponibile in quel momento a parlare per trovare soluzioni per i cittadini. Quindi è doveroso per me ricordare in quest'Aula Bruno Astorre e sono onorato di poterlo fare fare io a nome di tutto il Gruppo Lega. La tragica scomparsa di Bruno pone tutti noi davanti a un mistero dell'esistenza; soprattutto ci ricorda come ognuno di noi sia fragile nonostante l'apparenza di una vita agiata e di successo. Forse è questo il messaggio più profondo che Bruno lascia a tutti noi e che ci invita a guardare più in là, a vedere dentro gli occhi delle persone quella fragilità che ha ciascuno di noi, per farcene carico. È in fondo anche questo uno dei sensi più profondi della Pasqua che si avvicina. Bruno manca a tutti noi. Ci manca il riecheggiare della sua voce in *buvette*, ci manca la sua arguzia politica, ci mancano i suoi modi di dire, come quel "mannaggia li pescetti", che era solito pronunciare spesso, quasi a rimarcare orgoglioso le sue origini di provincia. Le migliaia di persone alle esequie nella sua Colonna testimoniano l'affetto e la stima incondizionata di tante persone che lo hanno conosciuto: parenti, amici, compagni di partito, certo, ma anche concittadini, avversari politici, persone comuni. Una stima frutto del suo appassionato radicamento territoriale, che ne ha fatto le sue fortune politiche. Bruno Astorre era un politico di razza; la politica l'ha appresa da ragazzo con Lavagnini, di cui è diventato il naturale successore, e l'ha praticata in tutta la sua vita. Sappiamo che per fare politica servono alcune caratteristiche: lungimiranza, altruismo, cultura, sensibilità, studio, ma anche scaltrezza, resistenza, pazienza, capacità di ascolto. Bruno le aveva decisamente tutte, pronto a difendere sempre gli interessi del suo territorio, il Lazio, e dei suoi cittadini. Affidabile, appassionato con gli amici, a volte implacabile con gli avversari, interni ed esterni. Credetemi, io ne so qualcosa, essendomi scontrato numerose volte con Bruno, che aveva il pregio di distinguere tra le questioni politiche e quelle personali, senza mai mischiare i due piani. Ne sono testimonianza le profonde amicizie che aveva con numerosi avversari politici - me compreso - che oggi ne piangono la scomparsa. Con Bruno Astorre questa Assemblea e il Lazio perdono un politico di serie A, ma soprattutto un uomo che con la sua giovialità e il suo umorismo ha saputo accattivarsi le simpatie di tutti noi, nascondendo a tutti noi il suo male di vivere. Ciao Bruno, in bocca al lupo. Ringrazio tutti voi per gli interventi appassionati. Abbraccio ancora i familiari, a cui diamo un affettuoso saluto.

In primo luogo, il calendario della settimana corrente è integrato con la seduta di domani, alle ore 10, la quale prevede la discussione, dalla sede redigente, del disegno di legge sull'equo compenso, approvato dalla Camera dei deputati, le ratifiche di accordi internazionali e la risoluzione approvata dalla 3a Commissione permanente sui diritti delle donne in Iran, nonché, ove concluso dalla Commissione, dalla sede redigente, il documento istitutivo di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Giovedì 23 marzo si svolgeranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time* con la presenza dei Ministri degli affari esteri, dell'economia e per la famiglia. Le votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria, già previste per giovedì, sono rinviate al 13 aprile. La prossima settimana sarà riservata ai lavori delle Commissioni. Nella settimana dal 4 al 6 aprile saranno discussi il decreto-legge sul PNRR e, ove approvato dalla Camera dei deputati, il decreto-legge sulla cessione di crediti d'imposta. La settimana dall'11 al 14 aprile sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni, a condizione che siano conclusi i predetti decreti-legge. Nella settimana dal 18 al 20 aprile si discuteranno le questioni pregiudiziali sul decreto-legge immigrazione, nonché lo stesso decreto-legge nel merito, inoltre il decreto-legge in materia di protezione di persone provenienti dall'Ucraina, ove approvato dalla Camera dei deputati. Nella settimana dal 26 al 27 aprile sarà discusso il decreto-legge sugli strumenti finanziari in forma digitale. Giovedì 20 e giovedì 27 aprile si svolgeranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time.* Il calendario potrà essere integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento sulla delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, imprese, collegata alla manovra di finanza pubblica e con il Documento di economia e finanza 2023.

Signor Presidente, colleghi, oggi si celebrano tre cose: una splendida relazione del Presidente del Consiglio; la giornata

affascinante e meravigliosa, ma qualche volta terribile, ossia la Giornata mondiale delle persone con sindrome di Down. Quanti sono? Le cifre sono un po' ballerine. Diciamo che, ogni 1.200 bambini, nasce un bambino bellissimo con una sofferenza genetica, con gli occhietti un po' a mandorla, con tanta dolcezza tanta voglia di vivere. Però le cifre ballano perché tra le nascite e le persone con sindrome di Down in vita c'è una bella differenza,

che soffre soprattutto di eccessiva solitudine delle istituzioni - i bambini non nascono. Ma c'è la sofferenza psicologica e fisica della perdita di vita attraverso l'aborto, perché il bambino o la bambina con sindrome di Down, di tanti medici e tanta cultura - mi avvio alla conclusone ma vorrei parlare delle condizioni di vita di queste persone meravigliose - non vengono fatti nascere, si ritiene meglio che non nascano. Sono bambini che portano avanti, nella vita, quando è loro permesso, dolcezza, memoria e soprattutto amore infinito verso chi li accoglie. Ebbene, non permettiamo un olocausto non dichiarato. È chiaro che non proporrò mai legislazioni restrittive per la libertà della donna, ma vorrei parlare

danno esempi bellissimi di pazienza, tolleranza e amore, questo amore che noi non dimostriamo verso di loro sempre e in maniera concreta.